Onorevoli colleghi, la Conferenza dei Capigruppo, riunitasi questa mattina, ha approvato modifiche al calendario corrente e il nuovo calendario dei lavori fino al 9 luglio. Oggi pomeriggio il senatore Tomassini ricorderà la figura di Giovanni Valcavi, recentemente scomparso, già senatore nella X legislatura. Seguiranno gli interventi dei rappresentanti dei Gruppi per cinque minuti ciascuno. Resta stabilito che la settimana corrente sarà riservata all'esame dei due decreti-legge in scadenza: sullo spettacolo e attività culturali e in materia di immunità Stati esteri ed elezioni dei COMITES. A tal fine gli orari delle sedute sono stati prolungati già a partire dalla seduta pomeridiana di oggi, che si concluderà alle ore 21; domani l'Assemblea si riunirà dalle ore 9,30 alle ore 14 e dalle ore 16 alle ore 22. Per giovedì 17 giugno è prevista una sola seduta antimeridiana che peraltro, in relazione all'andamento dei lavori e sempre al fine di assicurare il voto finale dei due provvedimenti richiamati, potrà proseguire nel pomeriggio dopo una sospensione tra le ore 14 e le ore 15. Pertanto il sindacato ispettivo, già previsto per la seduta pomeridiana di giovedì prossimo, non avrà luogo. Tale calendario è stato predisposto al fine di consentire un'ampia discussione e il voto di tutti gli emendamenti presentati. Pertanto, ove si rendesse necessario, a una determinata ora della mattina di giovedì 17 giugno, la Presidenza procederà alle sole votazioni degli emendamenti residui, senza ulteriori interventi. Come già stabilito, la prossima settimana sarà riservata ai lavori delle Commissioni, con particolare riguardo al decreto-legge sulla manovra economica. Il provvedimento sarà incardinato in Assemblea nella seduta antimeridiana di giovedì 1° luglio. La discussione generale proseguirà nel pomeriggio, fino alle ore 22 e, se necessario, nella seduta antimeridiana del giorno successivo. La ripartizione dei tempi di esame del provvedimento sarà stabilita anche in relazione al numero degli emendamenti, che dovranno essere presentati entro le ore 17 di mercoledì 30 giugno. Giovedì 1° luglio, alle ore 9, è convocato il Parlamento in seduta comune per 1'elezione di otto componenti del Consiglio superiore della magistratura. Voteranno per primi i senatori. Pertanto, la seduta antimeridiana dell'Assemblea avrà inizio alle ore 10,30. Le repliche dei relatori e del Governo sul decreto-legge relativo alla manovra economica avranno luogo nella seduta antimeridiana di martedì 6 luglio. Le sedute dì tale settimana, fino alla mattina di venerdì 9 luglio, saranno riservate alla discussione degli emendamenti. Infine, per quanto riguarda la sospensione dei lavori per le ferie estive, i Capigruppo hanno unanimemente convenuto sull'opportunità di tenere seduta nei primi giorni di agosto, a partire da lunedì 2.

Signor Presidente, onorevoli rappresentanti del Governo, onorevoli colleghi, ringrazio la Presidenza del Senato che mi consente la possibilità e l'onore di parlare del senatore Giovanni Valcavi che, scomparso da poco più di un mese, ha fatto parte, anni fa, della nostra Assemblea, ma ha soprattutto lasciato nel corso della sua vita, che ha attraversato un periodo storico molto significativo per la nostra Nazione, una traccia duratura alla comunità locale e a tutti noi, fondata su eterni valori etici, culturali, sociali e politici. Colgo l'occasione anche per salutare la moglie, il fratello e altri congiunti che sono presenti in tribuna e ci ascoltano. Giovanni Valcavi nasce a Desenzano del Garda nel 1926, ma ben presto si trasferisce in Lombardia a Varese e, in un arco storico che va dal 1940 ai giorni nostri, si segnala per impegno civile, professionale, politico e sociale. Ancora adolescente, convinto assertore del socialismo, di cui si è sempre dichiarato appartenente, si è schierato con le forze della Resistenza. Divenuto poi avvocato e soprattutto studioso di leggi, è stato fiduciario di importanti famiglie ed imprese: i Rotschild, i Borghi, i Gucci, ma anche gli operai e i dipendenti del calzaturificio di Varese e gli impiegati della banca sono stati da lui assistiti e sostenuti in numerose vertenze. Ha ricoperto il ruolo di Presidente in varie istituzioni pubbliche, quali l'ospedale di Varese, istituti bancari ed altro. Politicamente, per anni è stato eletto alla Provincia di Varese, e nel 1991 è stato eletto nel nostro Senato. Il percorso in Senato fu breve perché, nell'incompatibilità del ruolo parlamentare con quello di presidente della Banca di Luino, optò per il secondo, ma durante la presenza al Senato presentò ben 21 disegni di legge ed oltre 46 atti di sindacato ispettivo, mettendosi in evidenza per la sua lungimiranza ed esperienza. Patrimoni fondamentali che lascia a noi tutti sono quelli di aver fondato l'Università di Varese, di aver intrapreso numerose attività ed investimenti di solidarietà in Bolivia, di aver attivato una fondazione di studi giuridici che porta il suo nome e che ancora oggi viene visitata da studiosi di tutto il mondo, i quali hanno superato numericamente il milione. Per me, è sempre stata una personalità esemplare da imitare e seguire. Da quando sono stato eletto la prima volta mi ha onorato del suo affetto, della sua confidenza e della sua amicizia, guidando la mia opinione parlamentare, illuminandomi e fornendomi contributi che sono stati importantissimi per realizzare il disegno di legge sulla semplificazione del diritto societario, nella recente riforma del codice civile e, soprattutto, nella discussione e nel disegno di legge che reca modifiche al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria. Profondo e colto, ha mostrato sempre una passione civica ed umana, con tanto amore e sensibilità, in tante vicende pubbliche e individuali: valori che mi ha trasmesso e che ho cercato di imitare.

Ricordo quando mi informò di aver sposato Paola, mia valente collega ed amica: in quell'occasione il suo carattere scarno, burbero e ruvido si aprì in un sorriso con la felicità negli occhi. È stato sicuramente merito di Paola se è stato assistito amorevolmente fino all'ultimo minuto, continuando a donarmi e a donarci il suo prezioso consiglio. Concludendo, in sintesi, se dovessi esprimere la dote più importante di Giovanni Valcavi direi che è quella di essere proiettato nel futuro e quindi di essere attuale, moderno, anzi più moderno dei giovani. *(Applausi.

TONI *(IdV)*. Signor Presidente, colleghi senatori, rappresentanti del Governo, il Gruppo Italia dei Valori esprime il più sentito cordoglio alla famiglia per la scomparsa dell'avvocato Giovanni Valcavi, senatore della Repubblica nella X legislatura. Con lui scompare una figura di grande spessore umano, culturale, civile e politico, un uomo che ha attraversato l'intero Novecento, ricco delle sue idealità, profondendo la sua passione per gli studi giuridici dei quali è stato un autentico interprete. Si è spento lo scorso aprile, avendo vissuto sempre, con intensa passione e strenuo impegno, grandi battaglie; l'ultima, in qualità di presidente onorario del comitato organizzatore varesino - incarico che accettò rispondendo "obbedisco" quella per la rievocazione dei 150 anni dell'Unità di Italia, per lui un valore assoluto e intoccabile. *(Brusìo).* Presidente, neanche in una commemorazione si riesce ad avere un attimo di attenzione. Bresciano di nascita, varesino di adozione, da giovane studente si schiera per la libertà d'Italia contro la dittatura nazifascista, conosce Lelio Basso e aderisce al movimento socialista. Nei giorni difficili seguiti alla Liberazione rifiuta e condanna la violenza e la giustizia sommaria che pure a Varese, di cui sarà cittadino benemerito, non mancò. Quando il Partito socialista si riorganizza, nel secondo dopoguerra, non ha dubbi che debba essere una formazione pronta a rigettare qualsiasi dittatura, anche quella comunista. A Varese diventa un punto di riferimento della corrente riformista. La sua scelta socialdemocratica è l'unica possibilità di libertà e di liberazione dell'uomo dai condizionamenti economici, ma sempre all'interno di una società democratica. Si schiera con Saragat e con gli eredi del socialismo turatiano milanese, con Giuseppe Faravelli di «Critica Sociale». Quando si ricostruirà la storia del socialismo varesino del secondo dopoguerra si dovrà ricordare che Giovanni Valcavi è stato davvero l'esponente più autorevole del socialismo riformista, a Varese e non solo, erede di quella corrente che aveva profonde radici nella democrazia risorgimentale italiana. Nelle sue considerazioni, Garibaldi sarà sempre il grande protagonista delle battaglie per la libertà dei popoli, l'eroe - per lui - della libertà. Nel secondo dopoguerra le scelte di campo nella sinistra italiana e dentro lo stesso socialismo democratico non furono mai semplici. Pochi ricordano che all'interno dello stesso PSDI il pomo della discordia, come lo stesso Valcavi ebbe a scrivere, era l'adesione del Paese al Patto atlantico. Una sola delle tre correnti del PSDI era decisamente atlantista e Valcavi a Varese rappresentava una via mediana, che tentava di avvalorare scelte autonome dell'Italia. Aveva un'idea precisa della funzione dei partiti e della loro azione politica. Le correnti politiche nei partiti erano per Valcavi gli strumenti per l'esercizio della battaglia delle idee, per testimoniare libere scelte in campo politico. Giunse a coronare la sua storia politica con l'ingresso nel Senato della Repubblica, qui in quest'Aula, nella X legislatura, dove, come già ricordato, pur rimanendo per un breve periodo svolse un lavoro intenso ed impegnativo,

ma non rinunciò mai ad essere quello che aveva sempre voluto, liberamente, tornò alla sua professione ed ai suoi interessi culturali. Tra i tanti incarichi di prestigio, fu amministratore della Banca popolare di Milano, della Banca Rothschild e della Confederazione delle banche popolari. Ma Varese lo ricorda soprattutto come presidente della Banca popolare di Luino e Varese, come presidente dell'ospedale e come uno dei padri fondatori - tengo a sottolinearlo - dell'Università dell'Insubria, per il cui sostegno aveva creato anche la Fondazione Valcavi. Allievo dei professori Betti, Trabucchi ed Allorio, appassionato studioso di diritto, è stato autore di numerosi ed approfonditi scritti di diritto e di procedura civile, nonché di diritto fallimentare sulle maggiori riviste di settore. La sua sensibilità verso il prossimo lo porta ad impegnarsi in iniziative di beneficenza in Bolivia attraverso la donazione di attrezzature ospedaliere, ricoveri per anziani, asili, scuole e case per i contadini, dimostrando una particolare attenzione per i più deboli e per gli emarginati. Vorrei concludere con una mia riflessione. Credo che tocchi a noi oggi in quest'Aula far nostro il messaggio che Valcavi ci ha trasmesso: il senso pieno di un impegno, una vita al servizio del bene comune. scompare un uomo del Novecento che ha saputo affacciarsi al davanzale del terzo millennio carico forse solo della sua grande, intensa e ricca umanità.

Voglio ricordare Giovanni Valcavi come collega senatore della X legislatura, come uomo di cultura e di grande professionalità e impegno per la collettività. Come ha già ricordato il presidente Tomassini, Giovanni Valcavi ha svolto un lavoro rilevante in Senato: fece parte della Commissione sanità, dove ha dato un importante contributo impegnando tutta la sua preparazione, professionalità ed esperienza in campo sanitario e ospedaliero. Egli ha partecipato attivamente anche ai lavori alla Commissione giustizia, impegnandosi incessantemente nell'analisi delle problematiche e delle prospettive di riforma del processo civile, presentando sull'argomento anche diversi disegni di legge; il che lo portò ad essere chiamato a far parte della Commissione ministeriale per la riforma del codice di procedura civile. Grande merito gli si riconosce per il suo impegno intellettuale rivolto alla formazione professionale dei giovani e alla ricerca e allo sviluppo, tant'è che fu l'animatore e tenace realizzatore della nascita dell'Università dell'Insubria con sede a Varese e Como. Tutta la sua dedizione ed il suo impegno appassionato al servizio autentico della comunità si appalesa nella costituzione, attivata personalmente, della Fondazione Giovanni Valcavi, con lo scopo di favorire il finanziamento, lo sviluppo e la valorizzazione dell'attività di ricerca scientifica e tecnologica e di formazione ed aggiornamento professionale dei giovani, compresa la divulgazione e l'approfondimento di temi e questioni di carattere giuridico. L'avvocato Giovanni Valcavi fu un importante giurista di fama internazionale: a lui dobbiamo tutto il nostro riconoscimento e un sincero grazie per il suo operato.

e la lettura di una biografia è un'avventura nel tempo: date, avvenimenti, costruzioni.

non so se conoscessero in qualche modo la storia di quell'università, che per le cronache - è stata istituita il 14 luglio del 1998, quasi 12 anni (sta entrando nell'adolescenza). Era però dal 1972 che Giovanni Valcavi si batteva con tenacia e volontà straordinaria per portare nel suo territorio il luogo della formazione. Lo ha raccontato in un suo libro, di 30 capitoli, in cui c'è la storia dei

Poi vi è riuscito, però, e credo che questo sia il segno vero di un'attenzione straordinaria. Il logo dell'università è la stilizzazione di due fiumi che alimentano un corso centrale che divide, e insieme unisce, i territori del Varesotto

Successivamente, si laurea in legge all'Università statale di Milano. Nel periodo di frequentazione del liceo ha militato nella FUCI, l'associazione degli universitari cattolici,

Personaggio dalle mille sfaccettature, egli divenne un grande esperto di diritto; fu autore di numerosi scritti di diritto amministrativo, di procedura civile e di diritto fallimentare; divenne, tra l'altro, componente della Commissione ministeriale per la riforma del codice di procedura civile, presidente dell'ospedale di Varese, amministratore, per diversi anni, della Banca popolare di Milano e presidente della Banca popolare di Luino e Varese. A Varese si è prodigato per la nascita dell'Università Insubria dal 1972, con il supporto dell'allora sindaco di Varese, Mario Ossola e del presidente della Provincia, Fausto Franchi, istituendo nel 1975 la Fondazione studi giuridici avvocato Giovanni Valcavi, con propri adeguati capitali - questo non può che fargli onore - avente lo scopo di promuovere corsi professionali di specializzazione e di aggiornamento per gli avvocati.

a condividere i viaggi e le sedute del Senato con il senatore Bossi.

a volte pareva che non ascoltasse e che stesse pensando ad altro; invece raccoglieva tutto e le sue risposte erano di tutto rispetto.

con monsignor Pigionatti e don Manzoni al collegio De Filippi, senza dimenticare monsignor Pasquale Macchi, segretario particolare di Papa Paolo VI. Paolo VI. A conferma del suo credo l'elargizione di donazioni a favore dei tanti bisognosi: molte sono le testimonianze dei suoi aiuti a Nazareth e in Bolivia per la realizzazione di ospedali, ricoveri per anziani, asili e scuole. Per ultima, ma non ultima, la passione per la sua Varese, la divulgazione del dialetto, assumendosi l'onere economico della pubblicazione di poesie e vocabolario o meglio del «parolario bosino», ritenendo il dialetto una cultura antica. Infatti, quando ci incontravamo, parlavamo in varesino, in bosino. In un libro «Ricordi, vita professionale e pubblica per il diritto e per Varese», scritto dello stesso Valcavi, all'ultima pagina, nelle considerazioni sui valori perseguiti, si riconoscevano la sua grandezza ed umiltà. L'autore di queste pagine ha costantemente cercato di ispirare la sua condotta ed il suo operato, dove ha potuto, a quei valori che danno - a suo avviso - un senso alla vita, come la trasparenza del comportamento, il rispetto delle leggi e l'impegno ad assistere i clienti che hanno ragioni da tutelare e non hanno sempre i mezzi necessari, adattandosi anche alle loro condizioni economiche.

quando si è chiamati a commemorare qualcuno - nella fattispecie la figura di un concittadino, illustre e benemerito, come Giovanni Valcavi - e a ripercorrerne la sua biografia, mi chiedo sempre da che cosa si possa giudicare l'esistenza di un uomo. Si può dire in realtà come sia stato, annoverare le cose fatte, ma diverse possono essere le strade per giungere alla verità della sua vita. Nella sua breve, e pure intensa, partecipazione in quest'Aula, c'è da sottolineare quella passione che lo portò ad analizzare e suggerire, dall'interno di un'esperienza sviluppatasi nell'ambito dell'avvocatura ma non solo, problemi e prospettive relativi alla riforma del processo civile, come è stato già ricordato. In epoca di insistiti microregionalismi risorgenti e di steccati e separatismi, credo sia significativo ed opportuno rammentare l'impegno profuso da Valcavi per le tre edizioni del Vocabolario Bosino, in lingua dialettale varesina, segno di filologia affettiva

prossimi a una frontiera storica prim'ancora che geografica, segnata per entrambi dall'attrazione di un lago: Valcavi era nato a Desenzano del Garda, mio padre a Luino, che si affaccia sulla sponda lombarda del lago Maggiore; generazionale - intendo - di chi si trovò non ancora ventenne ad osservare, da dietro i vetri, in agguato, la campagna dell'infanzia ove sfilavano treni fra campi che improvvisamente vedeva trasformarsi nell'incendio della guerra. Del 1926 era anche Pietro Scoppola, a testimonianza di quei nostri padri (biologici e spirituali) che hanno attraversato le aspirazioni e le sconfitte di una generazione di laici e di credenti, fra resistenza e resa: di chi si è appassionato alla politica in modo non strumentale - come un mezzo, cioè, per conseguire un fine diverso dalla politica stessa ma come politica in sé, disegno per il futuro; come valutazione razionale del possibile e come sofferenza per l'impossibile; come chiamata ideale dei cittadini a nuovi traguardi; come tensione verso un'uguaglianza irrealizzabile e, come tale, tanto più perseguita ed agognata. Rammentare la figura di Giovanni Valcavi, oggi in quest'Aula, ha per me soprattutto questo significato: pensare ad una generazione che si è interessata alla politica più per quello che non riesce ad essere, piuttosto che per quello che è; un interesse quindi non per la politica in sé, ma per quel prezioso e insostituibile strumento in grado di muovere, modellare ed accrescere quella comunità che Valcavi ha servito con dedizione fino alla fine dei suoi giorni.

onorevoli colleghi, a conclusione di questo momento commemorativo non vorrei ripercorre altri episodi della vita di Giovanni Valcavi, che ne hanno segnato l'impegno civile e politico profuso per molti anni. Chi mi ha preceduto, infatti, è stato prodigo di ricordi e di particolari, spesso personali. Vorrei ricordare, invece, l'uomo e il politico prima ancora che l'avvocato o il senatore. Vorrei ricordarne, cioè, la cultura, intesa nell'accezione più ampia, la quale lo ha contraddistinto lungo tutto l'arco della vita: la cifra della sua testimonianza in ambito politico, professionale e privato che, in fondo, è il *fil rouge* che collega gli interventi finora svolti É una testimonianza complessa e a volte, apparentemente, contraddittoria. Quella politica si inserisce nel filone del socialismo riformista, cui approdò grazie all'incontro e all'amicizia con gli autorevoli eredi della concezione dell'uomo e della società di Filippo Turati. il riformismo milanese, ma anche quel socialismo di laici e di credenti sviluppatosi nel primo processo di industrializzazione ai piedi delle montagne del Nord Italia, in Lombardia come in Veneto o in Piemonte, fra cui - ad esempio - Francesco Forte, di cui fu amico, straordinaria figura di economista e socialista. Quella politica, che espresse sin dalla travagliata esperienza della costruzione del Partito socialista negli anni sul finire della seconda guerra mondiale e che proseguì con l'impegno nella società, iniziato con il lavoro nella Giunta provinciale di Varese e proseguito, sebbene avanti negli anni, con una breve ma intensa esperienza parlamentare. La profonda conoscenza del diritto monetario e bancario gli consentì di svolgere una variegata attività professionale: importante avvocato di diritto commerciale e finanziario; appassionato e raffinato studioso di questioni giuridiche, affrontate in scritti ancora oggi rilevanti; banchiere. Una definizione, quest'ultima, che forse non si addice completamente alla sua persona, almeno nell'accezione estrema, più in voga in questo periodo di crisi e che non ci fa ben pensare, ma l'impegno e l'interesse di Valcavi era diretto al settore bancario soprattutto per il suo impegno negli istituti di credito di tipo cooperativo. E ancora qua, la sua profonda radice nella cooperazione solidale e cristiana, come socialista, emergeva Fu infatti amministratore della Banca Popolare di Milano negli anni '60 e '70; fece parte per oltre un quinquennio nel Comitato direttivo della Confederazione mondiale delle banche popolari, delle quali difese con caparbietà, e a volte con intransigenza - un aspetto del suo carattere che potrebbe sembrare in contrasto con la riservatezza o la raffinatezza dei suoi gusti - la peculiarità, il principio della democrazia economica, secondo gli insegnamenti di Luigi Luzzatti. E lo ha fatto fino a poco tempo fa, nel 2008, quando, nel corso dell'assemblea della Banca Popolare di Milano ribadiva ciò che andava dicendo da qualche anno sui pericoli di quello che chiamava il gigantismo bancario, degli obiettivi mercantilistici e organizzativi, lontani dall'essenza del "fare banca", che avrebbero portato all'inevitabile crisi (così come si è poi verificato). Un'attenzione per gli aspetti "domestici" del mondo della finanza, che fa da *pendant* al suo modo di intendere, che emerge proprio da esperienze come quella del suo incarico al Senato, di cui ho parlato prima. Una vicenda che sembra uscita da un libro di Piero Chiara, che racconta, con sottile umorismo, storie argute e furbesche, ma bonarie, di provincia, fra Luino, Varese e Busto Arsizio. Chi ha avuto modo di essere in Senato durante il suo breve mandato ne ricorda l'assidua frequentazione delle sedute di Aula e Commissione, la presenza pressocchè costante in Senato. Presidente della Banca di Luino e di Varese, viene proclamato senatore nel marzo 1991, ma sapeva di optare a breve per la "sua" banca. Tuttavia, il titolo di senatore gli piaceva, non ci voleva rinunciare, era un coronamento della sua carriera. Non tanto e non certo per l'indennità (irrisoria rispetto ai suoi guadagni professionali), professionali), quanto piuttosto per il ruolo e il suo prestigio che però voleva conquistare, meritare il più possibile. Spero che questo breve ricordo, insieme a quelli precedenti, sia riuscito a rappresentare quella internazionalità di provincia

presentato dal Governo e giunto all'esame dell'Assemblea, converte in legge il decreto-legge 30 aprile 2010, n. 64, recante disposizioni urgenti in materia di spettacolo e attività culturali. Il provvedimento si configura come momento di singolare importanza e particolare rilievo politico cui questo ramo del Parlamento è chiamato a svolgere un'opera di riordino nonché ad affrontare e risolvere in maniera seria e coraggiosa i problemi che esistono all'interno di un settore fondamentale dello spettacolo: il comparto degli enti lirici. Nel ringraziare tutti i componenti della Commissione per il notevole livello di confronto svolto in discussione generale e per l'eccellente lavoro elaborato durante un lungo dibattito, desidero anche sottolineare la consistenza e il risalto dei molteplici e autorevoli interventi avvenuti in Commissione. da più decenni a questa parte, al settore della cultura, dello spettacolo e della musica. Bisogna risalire all'ormai lontano 1967 e precisamente alla legge n. 800 - la cosiddetta legge Corona, dal nome del ministro Achille Corona che la propose in Parlamento - la quale cercò per la prima volta di affrontare in modo sistematico e risolutivo una situazione quasi al collasso per la discontinuità e frammentarietà della legislazione precedente. La legge Corona, all'articolo 1, sostiene che «lo Stato considera l'attività lirica e concertistica di rilevante interesse generale, in quanto intesa a favorire la formazione musicale, culturale e sociale della collettività nazionale». Diciamo che il «Nuovo ordinamento degli enti lirici e delle attività musicali» forniva per la prima volta, con quella legge, una fotografia istituzionale del settore lirico-musicale, operando una classificazione tra enti di diverse dimensioni ed importanza, dalla quale sarebbe scaturito poi l'ammontare dei contributi pubblici. Tuttavia, va anche ricordato che in quel provvedimento, mentre viene confermato lo stato giuridico di ente autonomo lirico, viene ugualmente introdotto il concetto di «istituzione concertistica assimilata» in riferimento all'Accademia nazionale di Santa Cecilia e all'Istituzione dei concerti del Conservatorio Giovanni Pierluigi da Palestrina di Cagliari. Gli enti lirici allora erano 11, mentre le istituzioni concertistiche assimilate Ad essi venne attribuita personalità giuridica di diritto pubblico e gli enti furono sottoposti alla vigilanza del Ministero del turismo e dello spettacolo. L'articolo 5 della legge conferma che essi non hanno fini di lucro, assegnando loro come fine "la diffusione dell'arte musicale, la formazione professionale dei quadri artistici e l'educazione musicale della collettività". Dal punto di vista economico, il finanziamento statale fu svincolato dal gettito statale fu svincolato dal gettito erariale e stabilito nella cifra fissa annua di 12 miliardi. Nel contempo, si cercò di imporre alle amministrazioni degli enti il rigoroso rispetto del *budget*. Fu un fallimento totale poiché, se da una parte la concezione di finanziamento determinato in base a un ammontare fisso è in contrasto con l'esigenza crescente di capitali, dall'altra, le amministrazioni teatrali non si distinsero certo per oculatezza e rispetto dei vincoli di spesa. All'indomani, perciò, dell'entrata in vigore della legge n. 800, già una serie di provvedimenti tampone dovette far fronte alle emergenze di una situazione deficitaria gravissima, al punto che, nel 1984, lo stanziamento statale disposto è di ben 220 miliardi.

Si arriva, nel 1985, alla legge n. 163, che attraverso l'istituzione del FUS (Fondo unico per lo spettacolo) si propone di dare sistemazione definitiva ed organica agli interventi finanziari dello Stato a favore dello spettacolo nel suo complesso, per il presente e per il futuro. È chiamata anche "legge madre", poiché avrebbe dovuto preannunciare le future leggi di riforma del singolo settore. Certezza, predeterminazione, indicizzazione sarebbero state garantite attraverso un adeguamento triennale, da approvare in sede di legge finanziaria. Ma anche in questa nuova versione normativa la legge da pochi frutti. L'adeguamento viene difatti rispettato solo per i primi 4 anni. Negli anni '80 e '90 continua drammaticamente il processo di depauperamento di valore reale del FUS. Inoltre una serie di prescrizioni rigide e di lacune legislative incidono sempre più negativamente ed incagliano l'attività degli enti lirico-sinfonici. La forza lavoro occupata negli enti lirici, a volte eccessiva, mostra i tratti tipici del pubblico impiego, mentre i grandi nomi del circuito internazionale ricevono compensi altissimi, spesso al di fuori dalle logiche di mercato. Produzioni di grande rilevanza culturale sono rappresentate solo poche volte e i costosi allestimenti, ben lungi dall'ammortizzare il proprio costo, finiscono ad ammuffire nei depositi dei teatri. Il nodo fondamentale resta quello del finanziamento, sempre insufficiente - è vero - e collegato ad uno stato di emergenza permanente, che induce lo Stato a finanziare sempre e comunque gli enti, non discriminando - purtroppo, dico io - tra quelli che cercano una loro produttività e quelli che agiscono prescindendo del tutto da criteri di economicità. È in questo contesto di crisi che nella seconda metà degli anni '90 lievita e matura l'esigenza di un riordino e di una riforma degli enti lirici. Il decreto-legge n. 367 del 1996, prevede infatti la trasformazione dei 14 enti lirici pubblici, disciplinati dalla legge Corona, in altrettante fondazioni di diritto privato, il cui obiettivo, determinato dal legislatore, è quello di perseguire, senza scopo di lucro, "la diffusione dell'arte, la formazione professionale dei quadri artistici e l'educazione musicale della collettività". Tale trasformazione normativamente intervenuta e realizzatasi entro tre anni dall'entrata in vigore del decreto, ha prodotto una serie di modifiche estremamente complesse: oltre alla privatizzazione della veste giuridica, è subentrata una semplificazione del regime organizzativo, la privatizzazione del rapporto di lavoro, una razionalizzazione dei sistemi gestionali secondo criteri squisitamente aziendalistici. Ma, dal punto di vista dei costi e dei bilanci, poco però è cambiato. È noto a tutti, difatti, che le Fondazioni lirico-sinfoniche attraversano una fase di crisi dovuta alla crescita esponenziale della spesa per il personale. In particolare, a fronte di finanziamenti statali, sostanzialmente invariati dal 2003 ad oggi (pari sempre a circa 230 milioni di euro), la spesa per la contrattazione ha conosciuto un'impennata dopo l'abrogazione della norma calmieratrice di cui il sottoscritto era stato proponente nel decreto-legge n. 7 del 2005. Ebbene, proprio l'esplosione dei costi, dopo l'abrogazione di quella norma, testimonia l'urgenza di intervenire per riportare la spesa sotto controllo ed avviare procedure di risanamento idonee, pena il definitivo fallimento del sistema lirico-sinfonico italiano. Ecco, è questo - ritengo - lo spirito del decreto-legge È infatti intollerabile, onorevoli colleghi, che il contratto nazionale - non a caso fermo al 2003 - finisca per regolare aspetti solo marginali, mentre la sostanza della contrattazione avviene, nella maggior parte dei casi, a livello integrativo. Signor Presidente, è inconcepibile che il contratto collettivo sia una parte ben misera dello stipendio di queste maestranze. Pensi che il contratto integrativo raggiunge anche il 60 per cento di quello collettivo. Non può chiamarsi integrativo. E ciò perché i contratti integrativi prevedono indennità molto vantaggiose e remunerative. Quale è allora la filosofia del decreto? Il provvedimento normativa in oggetto riorganizza la struttura del contratto collettivo nazionale, attribuendo un importante ruolo di consulenza all'ARAN, in considerazione del carattere a tutti gli effetti di diritto pubblico delle Fondazioni lirico-sinfoniche i cui bilanci - ricordo a tutti - sono per la maggior parte finanziati da soggetti pubblici, non solo statali ma anche regionali, provinciali e comunali. cosa occorre per superare lo stallo che dura ormai da più di otto anni? Occorre innanzitutto che le parti contraenti siano indotte a firmare il prima possibile il nuovo contratto nazionale e, in secondo luogo, circoscrivere la stipula di contratti integrativi a particolari situazioni di impellenza ed emergenza. E difatti, a tal fine, il decreto ha introdotto il taglio del 50 per cento del trattamento economico aggiuntivo, qualora - solo qualora - il nuovo contratto non sia firmato entro un anno. Del resto, la firma del contratto collettivo consente il recupero rispetto a molti dei tagli e rappresenta dunque l'obiettivo principale verso cui tendere tutti gli sforzi. Una riflessione a parte merita la riproposizione delle norme sul blocco del *turnover*, le quali, ad onor del vero, sono state le uniche in passato a determinare un certo raffreddamento della spesa per il personale. Ho avuto modo di menzionare in Commissione alcuni fenomeni degenerativi, tali per cui non tutto il personale di ruolo svolgeva effettivamente i compiti per i quali era stato assunto. Sempre in materia di personale, sottolineo positivamente e vedo con favore la possibilità attribuita alle Fondazioni di ricorrere alle diverse tipologie contrattuali flessibili della cosiddetta legge Biagi, onde evitare la consueta trasformazione dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato per via giurisdizionale a seguito di massicci ricorsi alla magistratura. Vorrei infine ridimensionare il focolaio di polemiche esploso in questi giorni secondo cui nel decreto-legge figurerebbero distinzioni tra Fondazioni cosiddette di serie A e di serie B. Il decreto-legge non prevede alcuna distinzione fra Fondazioni, ai fini della concessione dell'autonomia. Appare tuttavia evidente la circostanza che ciascuna delle 14 Fondazioni lirico-sinfoniche riconosciute dallo Stato ha un proprio profilo, una propria storia, una propria tradizione per cui si caratterizzano in modo diverso in termini di gestione, ricavi, sostegno privato, radicamento sul territorio. A titolo di esempio, signor Presidente, voglio ricordare che il Teatro alla Scala di Milano destina solo il 50 per cento del suo bilancio al personale, a fronte di una media dell'80 per cento degli altri teatri. Lo stesso riceve un sostegno da parte dei privati pari al 50 per cento del suo bilancio e incassa dalla bigliettazione oltre il 20 per cento a fronte dì una media degli altri assai più bassa. La principale voce di spesa resta, comunque, il costo del personale, che ormai neppure il complesso dei finanziamenti dello Stato è in grado di coprire. Nel migliore dei casi, secondo gli ultimi dati disponibili del 2008, i fondi pubblici sono arrivati a colmare l'80 per cento di queste spese vive. Anche per quanto riguarda i contributi dai privati, in pochi hanno saputo sfruttare quel meccanismo di reperimento di fondi sul mercato, che era alla base della legge di riforma del 1998. La Scala mostra di essere un'eccezione, con i suoi 15 milioni raccolti nel 2008 (contro i 10 milioni di euro concessi dagli enti locali di Comune, Provincia e Regione e i 37,2 milioni di euro dello Stato). Buona anche la situazione di Santa Cecilia e quella del San Carlo. Quale deve essere allora l'obiettivo primario in sede di conversione in legge del presente decreto-legge? Direi innanzitutto quello di produrre un immediato e urgente intervento volto a riformare, negli assetti fondamentali, un settore in profonda crisi come quello dello spettacolo ed in particolare il settore lirico-sinfonico, tenendo conto, peraltro, delle più recenti istanze formulate in tale ambito anche dall'Associazione nazionale delle fondazioni lirico-sinfoniche (ANFOLS). E ciò al fine di razionalizzare in modo migliore le spese degli enti lirici e nel contempo implementare, oltre alla produttività del settore, i livelli di qualità delle produzioni offerte. La necessità e l'urgenza, dunque, della riforma sono ormai indeclinabili. Invocata per il settore lirico-sinfonico dagli stessi amministratori degli enti lirici, nonché dai medesimi lavoratori, si è resa non più procrastinabile dalla difficile situazione in cui versano molte delle 14 fondazioni lirico-sinfoniche del nostro Paese, dovuta alle consistenti spese di mantenimento di tali enti ed in particolare alle spese per il personale (circa 5.500 unità) che assorbono il 70 per cento del finanziamento pubblico. Per rendersi conto dello stato di crisi del settore lirico-sinfonico basti considerare che, ad oggi, la spesa per il personale sostenuta dagli enti lirici assorbe un valore economico superiore al finanziamento statale. Nel 2008,

a causa del continuo ricorso al credito bancario e nonostante la tempestività dell'erogazione dei contributi da parte dello Stato. Il presente decreto-legge reca, infine, disposizioni che riformano l'età pensionabile dei ballerini e dei tersicorei per i quali l'età di pensione, europei, viene portata a 45 anni di età. La nuova normativa sul pensionamento consentirà un risparmio di oltre 10 milioni di euro. Si tratta, del resto, di una disposizione in linea con gli ordinamenti stranieri e che consente una razionalizzazione opportuna della spesa. E comunque, viste le perplessità emerse in Commissione sull'ipotesi di mancata stipula del contratto collettivo nazionale, nonché sul blocco del *turnover*, ho comunque, in accordo con il Governo, più volte dichiarato la disponibilità a valutare positivamente emendamenti da parte di tutte le forze politiche che ne moderino la portata degli effetti, a condizione però di non perdere di vista l'obiettivo finale che il decreto-legge si prefigge: vale a dire, quello di produrre un immediato e urgente intervento volto a riformare, negli assetti fondamentali, un settore in profonda crisi come quello dello spettacolo e, in particolare, del settore lirico-sinfonico. Abbiamo ritenuto, pertanto, in Commissione di intervenire in modo prioritario sulla riforma del settore lirico, condividendo in questo la proposta del ministro Bondi di disciplinare più efficacemente i contratti integrativi che, ribadisco, devono seguire e non precedere il contratto nazionale. L'articolo 6, in particolare, interviene per meglio disciplinare il diritto d'autore attraverso un sistema di pubblicità legale quale il registro presso la SIAE

(Istituto mutualistico artisti interpreti esecutori), che con un precedente provvedimento del 30 aprile 2009 il prefetto di Roma aveva dichiarato estinto definitivamente per motivata e constatata incapacità di raggiungere gli obiettivi statutari finalizzati alla tutela di questi artisti. Onorevoli colleghi, sappiamo che il momento è molto difficile, forse il meno idoneo per discutere di una riforma globale e complessiva degli enti lirici e dello spettacolo più in generale. Le risorse sono scarse, il presente incombe e nessuno può tirarsi fuori dalla necessità di compiere sacrifici. Tuttavia, è proprio oggi, in questa sede, che vanno assunte decisioni fondamentali. Bisogna perciò avere oggi il coraggio di scegliere quanta parte della nostra attenzione e quante delle nostre risorse vogliamo davvero destinare alla costruzione del futuro di questo Paese in termini di enti lirici, di spettacolo, di patrimonio storico culturale. E ciò, affinché il mondo dell'arte, della cultura e della musica mantenga quella centralità di partecipazione e di scelta che, istituendo un circolo virtuoso tra formazione, produzione ed espressione creativa, consenta al nostro Paese di affrontare da protagonista la continua sfida del cambiamento.

era ovvio immaginare, signor Ministro, che si partisse da quella risoluzione condivisa, che ottenne anche il consenso delle parti sociali. no! Il Governo ha scelto, anche questa volta, la strada della decretazione d'urgenza, benché la situazione delle fondazioni lirico sinfoniche risulti, per chi abbia dato una veloce lettura ai bilanci, assai migliore

però, anche ricordare che, quando cambia il sindaco in una città (e il caso di Roma è quello più eclatante), cambia anche il sovrintendente, cambiano quindi gli apparati ed è dunque ovvio che, magari, lievitino anche le spese.

Vi è un'altra considerazione, che va chiarita in Aula, prima di affrontare i testi. Si dice che la maggior parte del finanziamento pubblico è destinato al costo del lavoro. Tra l'altro, stiamo parlando di lavoro intellettuale e culturale. A cosa dovrebbe essere destinato il bilancio di un ente lirico? Non è una normale disquisizione in un tempo di crisi ,perché c'è in questo provvedimento un *surplus* polemico - fatemi dire, quasi una resa dei conti nei riguardi di un universo considerato, pur nell'era della conoscenza e dell'informazione, un luogo non omologato, non controllabile, persino un po' sovversivo, qua e là. Si guardi la brutalità dei tagli apportati in questi ultimi mesi all'intera filiera dei saperi, a cominciare dalla madre di tutti i tagli, il decreto n. 112 del luglio 2008, per procedere con il complesso delle scelte fatte dalla destra in questi due anni; quando proprio dalla lettura dei dati risulta - attenzione - che il costo del lavoro è diminuito negli ultimi cinque anni e l'orario non è - ministro Bondi, ricordo una sua intervista a «La Stampa» del 2008 - di 16 ore settimanali, bensì di 24.

con un compenso - si badi bene, attribuito al nuovo entrante a zero anzianità - superiore ad una prima parte dell'Opera di Roma al massimo dell'anzianità. Il costo del lavoro in Italia è inferiore a quello rilevabile in Insomma, perché allora questo decreto tanto sbagliato, assurdo e astorico, che confligge con una buona politica culturale e persino con il buon senso di una Italia che ha ancora una forte riconoscibilità nel mondo per la musica, l'opera, il cinema, il teatro, la danza, il balletto, mentre la lingua italiana miete successi persino clamorosi all'estero proprio per le arie d'opera? Come mai dunque, in un simile scenario, la scure si abbatte su tutti i luoghi formativi, anche sul Fondo unico per lo spettacolo, sui beni culturali, sull'editoria, sulla ricerca, sulla scuola, sull'università? Tutto questo, intrecciandosi al bavaglio messo sull'informazione: tagli e bavagli, potremmo dire. Insomma, si vuole impedire con questo decreto anche di cantare, oltreché di parlare, di conoscere. Ma, fuor di battuta, si sappia, cittadini del villaggio globale che amate la musica dal vivo, e quella italiana, magari, in particolare, che con un'altra norma di questo testo, concernente il taglio alle trasferte dei musicisti, diminuiranno i viaggi all'estero e le rappresentazioni. Quindi, forse, non sentirete più l'Aida, la Traviata, la Tosca, la Bohème, la Turandot. È un eccesso di zelo, signor Ministro, signor Sottosegretario? Sì, insieme drammatico e grottesco, che forse ha un'origine profonda: quella stessa che ha portato nell'ultima manovra economica a sciogliere d'ufficio l'Ente teatrale italiano e a tagliare della metà i contributi già esigui agli enti culturali e, di nuovo, il Fondo per l'editoria. In quello che viene chiamato il capitalismo cognitivo-informazionale, i beni immateriali - si badi bene - non sono meno importanti di quelli materiali. la conquista delle coscienze e dell'immaginario collettivo pare essere la vera posta in gioco della stagione che stiamo vivendo. E dunque si usano le armate mediatiche della televisione generalista, di cui grazie al famoso conflitto di interessi il Governo e la sua maggioranza hanno il predominio assoluto, per omologare il pensiero e trasformare i cittadini - questo è il tema - in mero pubblico, in un'*audience* indistinta da sollecitare con programmi e *format* studiati per abbassare i livelli di acculturazione e di capacità critica, mentre cultura e saperi sono la nuova linfa dell'era digitale. Di qui, dunque, la vostra volontà - forse velleità, ci auguriamo - di occupare in modo simbolicamente violento, tutt'altro che tranquillo, i territori troppo infedeli della conoscenza. Certo, è molto meno sovversivo far guardare ai cittadini «L'isola dei famosi» e far loro ammirare i nuovi semieroi della società postmediatica. Eppure, l'Italia avrebbe delle fortune e dei tesori che chiunque ci invidia. nomi straordinari ne cito solo alcuni: da Pollini al compianto Sinopoli, da Morricone ad Abbado, da Ughi a Muti, così apprezzati da essere un mito o una speranza per i giovani, dall'Europa al Venezuela; oppure Carla Fracci con i suoi strepitosi balletti, che non piacciono forse al sindaco di Roma; o ancora le rappresentazioni di Puccini, Rossini, Donizetti, Verdi e Bellini. Forse

Questo è un punto che tanto inquieta noi, ma che ha colpito anche la sensibilità del Presidente della Repubblica, che più di una volta ha richiamato la Carta costituzionale, che dedica uno specifico articolo alla cultura e che è garante di questa iniziativa per il rilancio dell'attività della ricerca e della conoscenza. Insomma, non vi piace il lavoro intellettuale, troppo irregolare, troppo lontano dal potere politico, economico e mediatico. Meglio diradarlo, condannando addetti ed orchestrali, spesso di prim'ordine, a un precariato eterno, o magari ad andarsene all'estero. Se non è così, signor Ministro, io per primo, e penso tutti noi, saremmo ben lieti di ammettere di avere sbagliato. Anzi,

alla centralizzazione della contrattazione c'entra davvero poco. Siamo pertanto i primi a dire che quel testo andrebbe rivisto, come sicuramente andrebbe aggiornata - e vi sono tante nostre ipotesi in materia - la legge n. 800 del 1967,

taglieggio proprio nei punti più importanti. Come mai? Spero che ce lo direte. Ma il nostro atteggiamento di forte contrarietà inizia persino dal titolo, assurdo e incongruo, di questo testo perché non riguarda affatto le attività culturali: è un testo di tagli e tutt'altro che di rilancio del settore.

sui punti essenziali ancora non vi è nulla di fatto. Sì, è stato tolto, per doveroso stralcio, l'articolo su Cinecittà, che proprio non c'entrava nulla; come pure è stato ottenuto qualche risultato dai nostri emendamenti, anche con il relatore: penso alla riduzione dal 50 al 5 per cento del contratto integrativo (c'è un emendamento che propone un taglio dell'1 all'anticipo a fine 2011 - un anno di meno - del bloccodel *turnover*, all'aumento dal 15 al 30 per cento delle possibili assunzioni a tempo determinato. I punti chiave però sono ancora lì, proprio a cominciare da quel combinato disposto degli articoli 2 e 3 che dà di questo decreto il senso e la chiave di interpretazione: tagli e tagli, blocco delle assunzioni, prepensionamento - che poi è quasi un licenziamento - per ballerini e tersicorei, commissariamento dell'istituto mutualistico attraverso il controllo di ben tre soggetti, tra Presidenza del Consiglio e Ministeri, l'unico punto che effettivamente meritava l'urgenza. conducendo una battaglia di opposizione qui in Aula, con più di 350 emendamenti, di cui tanti significativi, che sono stati discussi insieme alle organizzazioni sindacali e a tutte le associazioni riunite sotto la sigla "MovEm09". Andremo a fondo, perché non ci piace un cattivo senso comune. Ce lo insegnò Gramsci (lei, Ministro, cita ogni tanto qualche classico, e io gliene sono grato): proprio Gramsci ci ammoniva che un certo senso comune non va bene, e va rovesciato in un nuovo senso comune. Dobbiamo dire con molta nettezza che l'intervento pubblico, la vecchia idea del Novecento, oggi vuol dire un'altra cosa: valorizzazione dei beni comuni. Dobbiamo sapere che la cultura e la musica hanno un costo primario autorevole, che è stato sottolineato da tanti autori. Penso a qualche autore molto classico che certo piacerà a tanti di noi e voi, come Adorno, oppure, per chi ama il genere più moderno, moderno, alle frasi sulla musica e sulla sua importanza recitate a Woodstock da Jimmy Hendrix. Quell'armonia realizzata sul piano artistico di cui parlava Adorno deve sempre contenere ‑ diceva ‑ un un elemento di protesta nei confronti della realtà, una dimensione utopica, una promessa di felicità, secondo la definizione che lei sa, Ministro - egli traeva da Stendhal. E, tra le arti, proprio la musica è quella meno rappresentativa dell'immediatezza: è quella che, per fortuna, quella che ci fa sognare e immaginare un futuro più bello, che ci accompagna durante la nostra vita e ci fa anche sopportare i momenti più difficili. Del resto, nessuno dei *media*, per nuovo che sia, potrà fare a meno della musica. Guardate bene: la musica, unico fra i mezzi di comunicazione di massa, ha attraversato indenne 1.700 generazioni di linguaggi delle culture tribali e orali, 300 generazioni figlie della scrittura, e sta passando l'attuale era digitale con grande impulso, e l'era digitale è stata prefigurata proprio da alcuni grandi autori moderni, come John Cage o Luciano Berio. Ecco perché va sfatata l'idea iniqua, un po' penosa, che la produzione di musica o di baletto sia una spesa, e non un invece un investimento. Si chiede il Governo italiano, perché il Governo francese investe nella sola Opera di Parigi 105 milioni di euro? di minoranza*. Questo, a fronte di un Governo Berlusconi che per tutto il settore, (tutto: dall'opera, al teatro, alla musica, al cinema, alla danza agli spettacoli viaggianti) per il 2010 ha stanziato poco più di 400 milioni di euro, e per il 2011 ha previsto poco più di 300 milioni di euro? Sì, perché questo provvedimento si inquadra nei tagli, nelle riduzioni drastiche e inesorabili del Fondo unico per lo spettacolo, che è stato diminuito in pochi anni, da quando governava il centrosinistra, di tantissimi milioni di euro. E ancora, vorrei aggiungere

con l'investimento sulla cultura, la disoccupazione decrescesse del 25 per cento e, tra l'altro, si abbattesse il numero - il più alto in Europa - di tossicodipendenti.

pura e semplice a determinare le scelte nell'ambito culturale, ma una più complessa politica di economia della cultura, perché la politica culturale ha una sua specifica forma anche di politica economica, che non può essere uguale a quella di altri settori. La merce cultura non è come tutte le altre: è un luogo non solo di allocazione di risorse, ma anche di crescita morale e civile.

(gli emendamenti sono poi riassunti nel testo che consegno), che noi immaginiamo, signor Ministro, di andare presto ad una riforma di un settore così delicato. Ci sono stati tanti illustri personaggi che hanno anticipato la riforma; penso ad un sovrintendente che piacerà a tutti: Antonio Ghiringhelli, del Teatro alla Scala di Milano, che già negli anni '50 indicava delle linee interessanti. Penso che dovremmo fare presto, signor Ministro, perché a furia di tagliare - e spero che queste parole vengano prese nel verso giusto e amaro di chi le scrisse con grande autorevolezza,

Signor Presidente, la questione pregiudiziale che il Gruppo dell'Italia dei Valori ha presentato evidenzia diversi profili di illegittimità costituzionale,

Vorrei appuntare il mio intervento su uno degli aspetti che sono stati individuati sotto il profilo della illegittimità, e cioè quello della mancanza dei presupposti di necessità e di urgenza in questa materia.

I parametri indicati dagli articoli 76 e 77 della Costituzione...

trattati dalla Corte costituzionale con grande cautela, nel senso che la Corte vi ha fatto ricorso solo nei casi di violazioni assai gravi, preferendo non interferire nel profilo del circuito politico.

e della soggezione della giurisdizione e dell'amministrazione alla legge, l'adozione delle norme primarie spetta agli organi o all'organo il cui potere deriva direttamente dal popolo», ovvero alle Assemblee legislative. La attribuzione di poteri normativi al Governo, pertanto, ha «carattere derogatorio rispetto all'essenziale attribuzione al Parlamento della funzione di porre le norme primarie nell'ambito delle competenze dello Stato centrale».

secondo il dettato dell'articolo 77 non può essere sostenuta e utilizzata con semplici frasi di stile come, peraltro, leggiamo proprio nel caso del decreto-legge al nostro esame. Nella relazione introduttiva, infatti e come spesso capita nei decreti-legge, si usa una frase di stile in cui si dice che questa materia deve essere disciplinata per ragioni di necessità e urgenza. Si tratta evidentemente di una clausola di stile che non può legittimamente supportare l'utilizzo dello strumento del decreto‑legge, vieppiù in un caso come quello all'esame dell'Aula. Ricordo le trascrizioni degli interventi fatti in Commissione dal relatore Asciutti nella

Bondi, che la Commissione istruzione del Senato aveva ripetutamente chiesto e ottenuto un confronto con il ministro Bondi per discutere le linee del riordino del settore e che ciò era puntualmente avvenuto in ben tre audizioni:

denuncia ancora una volta l'utilizzo indebito dello strumento del decreto-legge e tecnicamente pone la questione pregiudiziale rinvenendo svariati profili di incostituzionalità.

Grazie,

signor Presidente: il 18 marzo 2009, più di un anno fa) ad un documento comune si concludeva con l'impegno ad affrontare il tema in termini termini legislativi all'interno di un confronto fattivo, al quale noi avevamo dato una disponibilità politica importante. Ciò evidenzia la dimensione della discussione e dell'approfondimento del tema in questione, a noi molto caro. C'era un tema di merito legato ai numeri e alla *governance* delle fondazioni lirico-sinfoniche, al loro approccio, al loro controllo, alla loro produttività e alla loro capacità di svolgere effettivamente il ruolo che la legge del 1996 aveva

È evidente che, per motivi diversi da quelli effettivamente esposti, il Governo ha deciso di procedere con questo tipo di

si provvede ad una nuova formula di delega, delegificando la materia; infatti si delega il Governo a provvedere ad una riforma tramite regolamenti ministeriali. Si tratta di un atto credo unico (forse il primo) e ingiustificato, che toglie al Parlamento la possibilità di intervenire con giudizio rispetto al provvedimento

si sia ancora in tempo a ritirare il provvedimento e a provvedere con un disegno di legge. Il Partito Democratico ha dato la propria disponibilità a seguire *iter* agevolati per arrivare ad una conclusione. Non vi è alcun motivo di urgenza e necessità, non vi è alcun motivo di delega al Governo a provvedere non con un atto legislativo, ma con regolamenti ministeriali. Credo che oggi sia un giorno triste: ho cominciato

Presidente, colleghi, con questa questione pregiudiziale di costituzionalità desideriamo chiedere, come senatori del Partito Democratico, di non procedere all'esame degli articoli del disegno di legge n. 2150, di conversione del decreto-legge n. 64 del 2010. Diverse disposizioni del disegno di legge generano, infatti, rilevanti perplessità sotto il profilo della legittimità costituzionale.

componenti del PDL della Commissione cultura, poche ore fa hanno rivolto un appello al Ministro, con il quale chiedono di modificare il decreto sulle fondazioni liriche e di scegliere la via del disegno di legge. Ci associamo, Ministro, a questa richiesta che - converrà - è un fatto politico.

la pesante ingerenza sulla contrattazione collettiva operata dal Governo. Innanzitutto, il taglio di una parte della retribuzione integrativa, operato mediante decreto-legge, è una disposizione senza precedenti. In secondo luogo, la previsione che il contratto collettivo nazionale di lavoro delle fondazioni lirico-sinfoniche sia sottoscritto da una delegazione datoriale avvalendosi della collaborazione dell'Agenzia per la rappresentanza negoziale nelle pubbliche amministrazioni (ARAN) e poi sottoposto al controllo della Corte dei conti appare del tutto incongrua, dato che non ci si trova di fronte ad enti pubblici. Queste norme, assieme al divieto di assunzione di personale amministrativo, artistico e tecnico, anche in adempimento di obblighi di legge, comportante aumenti del contingente numerico del personale, o al divieto di rinnovi dei rapporti di lavoro che, in base a disposizioni legislative o contrattuali, comporterebbero la trasformazione dei contratti a termine in contratti a tempo indeterminato, ledono fortemente l'autonomia delle fondazioni lirico-sinfoniche e violano manifestamente l'articolo 33, comma 6, della Costituzione, che assicura alle istituzioni di alta cultura, alle università e alle accademie il diritto di darsi ordinamenti autonomi. Il decreto, infine, disciplina minuziosamente la materia delle attività culturali, in contrasto con l'articolo 117, comma 3, della Costituzione per quanto riguarda la legislazione concorrente tra Stato e Regioni. In realtà, siamo di fronte all'ennesimo provvedimento centralista che non valorizza e mette sullo stesso piano le grandi peculiarità della storia del teatro italiano,

O è troppo poco liberale, o troppo lasciato all'autonomia degli enti, che i rimborsi siano determinati dai successi dei nostri teatri all'estero, come Stéphane Lissner, caro relatore Asciutti, le ha ricordato nell'audizione? L'autonomia dei sovrintendenti dei teatri è questa. O forse, Ministro, in piena sintonia con la manovra economica che stiamo esaminando, il suo ruolo è solo quello di rassicurare il manovratore Tremonti, relegando il sapere e la cultura italiana al luogo del saccheggio delle risorse? Riaffermando le ragioni di incostituzionalità, noi ribadiamo la disponibilità, già manifestata in Commissione, di approvare in poche ore, in sede deliberante, la parte riguardante l'IMAIE e di costruire un disegno di legge condiviso, da votare in un tempo stabilito, sulle orme di quella risoluzione sugli enti lirici approvata all'unanimità dalla 7 a Commissione con il suo consenso, ministro Bondi. È ancora d'accordo, signor Ministro, con quella risoluzione? Allora accetti, se è d'accordo con quella risoluzione, come propongono gli onorevoli Granata e Barbieri, di ritirare questo decreto-legge.

Signor Presidente, signor Ministro,

il grandissimo patrimonio culturale, musicale e civile rappresentato dalle fondazioni lirico-sinfoniche nel nostro Paese, se non avessimo un'idea grande e bella dell'Italia e la convinzione fortissima che l'Italia è la sua cultura (la sua cultura musicale, lirica, sinfonica, coreutica), è il suo teatro, il suo cinema, lo spettacolo e che lì è l'identità del nostro popolo che si esprime in ogni teatro, in ogni città, nella provincia italiana del Nord e del Sud; se non avessimo la convinzione che essa deve continuare nelle nuove generazioni e nel loro talento e che deve continuare ad essere luogo di attrazione per i giovani di ogni parte del mondo; se non ci sentissimo, come ci sentiamo, responsabili del rilancio del nostro Paese anche attraverso la salvezza della sua bellezza e la promozione della sua missione culturale e musicale nel mondo, nei teatri di tutto il mondo di Pechino, Nuova York, Buenos Aires - per costruire il futuro del mondo, della sua coscienza e della sua civiltà universale anche con la cultura e la musica del nostro Paese; se non fossimo consapevoli che lì si esprimono competenze, professionalità, ricchezza per il Paese; se non ci importasse di tutto questo, se non sentissimo, signor Ministro, molto forte l'allarme in noi e intorno a noi, oggi non chiederemmo, ai sensi dell'articolo 93 del Regolamento del Senato, di sospendere in Aula l'esame del provvedimento del suo provvedimento - che ci appare così povero, così inadeguato, così miope e dannoso rispetto alle sfide che ho ricordato. Siamo mossi, come hanno già detto i colleghi, dalla risoluzione approvata all'unanimità in 7a Commissione il 18 marzo 2009: da lì doveva sortire un disegno di legge. Ancora in queste ore si chiede, lo fa anche la Camera dei deputati, che ci si fermi e che ci si orienti su un disegno di legge. In quella risoluzione si indicavano obiettivi precisi: l'incremento delle risorse per il Fondo unico per lo spettacolo, il raccordo tra i diversi enti, la destinazione dei fondi per la qualità, il ruolo e il contributo degli enti locali, la responsabilità della gestione. Lì dovevamo rimanere; da lì dovevamo partire; lì dobbiamo tornare. Invece, tutto questo è stato messo da parte dal Governo, sostituito da un decreto che delega semplicemente il Ministro al riordino ordinamentale e organizzativo, nel segno puro del centralismo. Non definisce né la *governance* né la responsabilità gestionale; non incentiva i privati; impoverisce le fondazioni, i lavoratori, gli artisti, i nuovi talenti; non mette affatto gli enti lirici nella condizione di uscire dai problemi drammatici in cui si trovano: il rimedio è peggiore del male, come se si trattasse di poca cosa marginale nella vita del nostro Paese. Solo una forte volontà condivisa può portare alle giuste soluzioni in quest'area. l'arte, musica, la cultura in Italia non sono un settore tra i tanti: sono una questione vitale per la Nazione. Hanno a che fare con la sua libertà, con il nutrimento della coscienza civile. Dobbiamo sapere che il no alla cultura è un no alla libertà. Parliamo semplicemente, qui, oggi, della nostra Patria, del suo essere, della sua consistenza, del suo sentimento comune, di ciò che la fa riconoscere nel mondo. Ciascuno di noi qui rappresenta dei territori, rappresenta tutta l'Italia, ma anche tante parti diverse d'Italia, e sa dove stanno la mente e il cuore della nostra gente, non vede l'ora di poter assaporare la cultura, la musica, il teatro. Nessuno davvero può impedire questa visione, questo desiderio. Nessuno può restringere i confini di questa aspirazione nazionale. Fermiamoci: questo provvedimento non è all'altezza del compito. Non crede, signor Ministro, che la tradizione culturale italiana si attendesse ben altro? Non possono i tagli essere una politica, una riforma: sono semplicemente una rinuncia, sono una sconfitta, sono un danno. Concludo, signor Presidente, ricordando che 135 anni fa in quest'Aula, da poco inaugurata,

Giuseppe Verdi se ne usciva con questa semplice espressione: «Dote ai teatri. Dote ai teatri e non imposte». dote, è la parola appropriata, quella che evoca un'eredità da trasmettere per il futuro. Senza i teatri non ci sarebbe stata l'Italia unita, quell'Italia unita che anche Verdi aveva costruito perché non rimanesse - come disse povera, debole, senza libertà e semibarbara. Colleghi, conviene che sospendiamo l'esame di questo provvedimento, che ritorniamo alla comune risoluzione. Pensiamo insieme come dare forza vera, efficacia, trasparenza alle fondazioni lirico-sinfoniche, come dare vita all'Italia, *(Commenti dal Gruppo PdL).* Colleghi, fermiamoci! Non faccia il Governo, non faccia il Parlamento ulteriori danni a questa nostra Patria, già molto sofferente.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, desidero innanzitutto ringraziare

per il lavoro che, insieme, abbiamo svolto in queste ultime settimane. Questo provvedimento, infatti, giunge in Aula dopo

sono giustificate, a mio avviso, dalla gravità della situazione nel settore lirico-sinfonico del nostro Paese: una gravità che nessuno può ignorare e sottovalutare. Avevo annunciato la necessità di un decreto, senza considerarlo, però, come un provvedimento blindato, ma, al contrario, come un provvedimento - come come poi è avvenuto realmente - aperto al confronto in Parlamento. Infatti - e credo che anche i colleghi

Grazie,

alla normalità, sotto controllo, le condizioni innanzi tutto economico-finanziarie delle fondazioni lirico-sinfoniche nel nostro Paese.

nel nostro Paese. Sono convinto - l'ho detto anche durante il dibattito in Commissione - che nessuno ha il monopolio della difesa delle ragioni della cultura nel nostro Paese. Il Governo, la maggioranza che lo sostiene, chi vi parla in questo momento, che ha la responsabilità dell'importante Ministero dei beni e delle attività culturali, al pari dell'opposizione sentono acutamente il problema del ruolo che la cultura può svolgere, tanto più in un Paese come l'Italia in cui - come è stato ricordato da molti colleghi

Se si pensa però, senatore Vita, che questo decreto-legge si abbatta sulla lirica perché considereremmo la lirica come un comparto della cultura sospetto, penso che ciò voglia dire abdicare al buon senso e soprattutto abdicare, da parte dell'opposizione, ad un ruolo effettivamente di governo. Un ruolo di governo non ignora la realtà in cui si trova la cultura oggi, e soprattutto non ignora, in particolare, le condizioni in cui si trova un settore della cultura particolare come quello lirico-sinfonico nel nostro Paese.

una realtà con la quale dobbiamo fare i conti e con la quale fanno i conti tutti i Governi in Europa, e lo dico senza alcun spirito polemico. Così come la crisi e le difficoltà del settore della lirica in Italia non le ho inventate io. Queste difficoltà non derivano soltanto dalla mancanza di risorse, di finanziamenti. Credo che la crisi ci costringa a rivedere il ruolo dello Stato nella cultura e soprattutto a ridurre innanzitutto

posso assicurarvi che il mio impegno è di salvaguardare gli istituti culturali, che rappresentano davvero un'eccellenza del nostro Paese, ai quali il nostro Paese non può rinunciare. Ma possiamo fare qualche sacrificio proprio per indirizzare le risorse che abbiamo a disposizione a favore degli istituti culturali più importanti, così come possiamo fare qualche sacrificio per quanto riguarda invece i finanziamenti a pioggia. la situazione in cui si trova il settore della lirica in Italia richiede riforme, interventi coraggiosi. Questa crisi è sotto gli occhi di tutti e non da oggi, da anni. Tutti sappiamo che questo settore si trova in una crisi difficile, che aveva ed ha bisogno di interventi e riforme coraggiosi. Ebbene, io mi sono assunto la responsabilità di proporre al Parlamento e al Paese una riforma che non intende scoraggiare questo settore e metterlo in difficoltà, ma intende salvare dal fallimento il settore della lirica sinfonica, nel nostro Paese. Questo è il mio intendimento e quello del Governo. Del resto, onorevoli senatori, ricordare alcune cifre di questa crisi, in modo che tutti ne siamo consapevoli. Nel 1996, una legge proposta dal Governo di centrosinistra, in particolare dall'onorevole Veltroni, privatizzò,

che tutti speravano, come oggi credo tutti possiamo riconoscere. Quali sono i dati fondamentali di questa crisi, di questa difficoltà del settore della lirica? Altrimenti, infatti, non si spiegherebbe la mia decisione di assumere e

A favore degli altri settori dello spettacolo sono indirizzati interventi minori: a favore del cinema noi spendiamo il 19 per cento del fondo unico dello spettacolo (90 milioni di euro); per la musica soltanto il 14 per cento; per la prosa soltanto il 16 per cento e per la danza, un settore altrettanto importante, soltanto il 2 per cento dei finanziamenti globali. Come vedete, c'è chiaramente uno squilibrio

l'Italia ha un'altra specificità. La nostra storia non è paragonabile a quella della Francia, perché noi abbiamo 14 fondazioni lirico-sinfoniche, diverse le une dalle altre,

il 60 per cento dai contributi dello Stato. Soltanto il 20 per cento delle entrate delle fondazioni derivano dal contributo degli enti locali,

dal contributo dei privati. A questa situazione, onorevoli senatori, deve aggiungersi il fatto che i debiti accumulati dalle fondazioni lirico-sinfoniche dal 1996 ad oggi ammontano ad oltre 300 milioni di euro. Il patrimonio iniziale dei vecchi enti lirici è stato praticamente azzerato. Per non parlare degli interventi straordinari che ogni anno sono necessari da parte del Ministero per i beni e le attività culturali per ripianare le perdite,

siamo davvero di fronte ad una crisi grave del settore che deriva da molte ragioni che non voglio qui ulteriormente approfondire. per concludere, che il decreto interviene su tutte queste questioni: dal sistema di contrattazione collettiva al sistema di assegnazione dei contributi pubblici, per il futuro, dalla riforma dei sistemi di gestione delle singole fondazioni lirico-sinfoniche fino all'adeguamento della disciplina italiana a quella europea in materia di trattamento previdenziale dei ballerini. Su questo spero sarà dato atto a me, al Governo, al Parlamento di aver affrontato e risolto una questione che nessuno prima d'ora aveva affrontato e risolto. Su tutti questi problemi, onorevoli senatori, il confronto, - lo ripeto - è stato costruttivo. Il testo è stato modificato profondamente in Commissione e credo che il testo che giunge in Aula sia migliore rispetto a quello che io e il Governo abbiamo presentato

garantire un futuro ad una delle tradizioni più illustri e più importanti della nostra cultura e del nostro passato.

far rilevare al Ministro che egli ha esposto il contenuto del provvedimento, ma non ha risposto alle obiezioni che erano state fatte sulle pregiudiziali di costituzionalità. Non ho sentito un argomento che abbia attinenza col tema sul quale noi fra poco voteremo. *(Applausi

Signor Presidente, colleghi, signor Ministro, lei sa bene che noi del Partito Democratico abbiamo svolto in Commissione un lavoro serio, responsabile, fattivo per contrastare questo decreto-legge e cercare di modificarlo per quanto possibile. Si tratta di un provvedimento che abbiamo giudicato sbagliato, dannoso per le fondazioni lirico-musicali, per il mondo dello spettacolo e della produzione culturale.

signor Presidente. Dicevo che abbiamo ritenuto doveroso contrastare questo decreto‑legge perché abbiamo a cuore le sorti della cultura italiana, coerentemente con i nostri valori, con i nostri principi civili, sociali politici. La cultura è un valore in sé; è un fattore di sviluppo civile, come hanno già ricordato i colleghi che mi hanno preceduta, ma è anche un fattore di sviluppo economico; favorisce la coesione sociale, in quanto costituisce l'elemento di maggiore identità dell'essere italiani oggi. Soprattutto la lirica costituisce un elemento di identificazione della nostra storia, della nostra tradizione, della nostra cultura, cultura, del nostro stare nel mondo, della nostra - vorrei dire - riconoscibilità nel mondo. Ma evidentemente non è questo il punto di vista del Governo e della maggioranza che lo sostiene. Ogni intervento sulla cultura è stato finora un colpo per renderla agonizzante, metterla in difficoltà, indurla a vivacchiare, ad arrangiarsi. Lo Stato si ritira, coadiuvato, devo dire, da una sempre più scadente programmazione televisiva, che abbassa il livello della conoscenza, di capacità reattiva, di senso critico dell'opinione pubblica. È meglio avere coscienze plagiate, acquiescenti. I contenuti di questo decreto sono una spia di un atteggiamento più generale del Governo verso la cultura. Mi dispiace che il ministro Bondi

addirittura un taglio a tutti gli istituti culturali, rientrato in parte soltanto grazie all'intervento, responsabile e saggio, del Capo dello Stato; la cancellazione con un colpo di spugna di enti di ricerca che svolgono spesso attività uniche nel loro genere; i tagli all'università, aggravati dalla manovra, che mettono in ginocchio le nostre università e la ricerca universitaria;

c'è un disegno che punta ad abbassare il livello di reattività critica dei cittadini e degli elettori. Anche per questo noi siamo contro questo decreto‑legge. Ma non sono poche anche le ragioni di merito che abbiamo discusso e presentato con grande consapevolezza e competenza, soprattutto da parte di alcuni membri della Commissione. Ci aspettavamo una riforma seria delle fondazioni lirico‑musicali, come avevamo proposto anche noi, come aveva proposto l'intera 7a Commissione, all'unanimità, e invece ci siamo trovati di fronte a un provvedimento tagliato con l'accetta - mi consenta, signor Presidente che contiene un paradosso già dal primo comma del primo articolo (una delega al Governo in un decreto-legge) e si limita a cancellare poi l'autonomia delle fondazioni, che è il loro punto di forza

Al posto dell'autonomia vi è questo burocratismo centralistico, che qualche volta rasenta l'autoritarismo: noi siamo allora per promuovere più qualità anche per le fondazioni lirico-musicali, per le istituzioni culturali e dello spettacolo, ma con questo decreto si avrà meno qualità e minore produttività. Certo, qualche miglioramento c'è stato, anche grazie alla nostra attività emendativa che è stata portata avanti con forza. Voglio ricordare in primo luogo lo stralcio dell'articolo 5, riguardo a Cinecittà: era assolutamente fuori luogo presentare un lungo articolo sul cinema quando proprio in Commissione abbiamo da tempo in discussione una legge sul cinema; su un testo. Invece nell'articolo 4 si interviene pesantemente proprio sullo

per i lavoratori dello spettacolo e delle fondazioni. Sono cambiati i tempi per il divieto di assunzione; certamente, si è migliorato qualcosa in merito al pensionamento dei ballerini. tuttavia un provvedimento che non promuove la produzione culturale e lirica ma la deprime; resta quell'impostazione centralistica e punitiva che noi abbiamo denunciato e tentato in tutti i modi di contrastare.

a chiacchierare con il senatore Cutrufo, che lo distrae continuamente. Mi dispiace, signor Sottosegretario, che lei sia qui a chiacchierare; è vero, ci ha ascoltato per molto tempo in Commissione, ma se lei viene in Aula è per ascoltare e non per chiacchierare. Dicevo che noi continuiamo a denunciare l'impostazione centralistica e punitiva di questo provvedimento e mi auguro che il Ministro e il Governo possano ripensarci e ritirarlo, come abbiamo chiesto sin dall'inizio. In ogni caso tenteremo anche in quest'Aula di continuare a migliorarlo.

purtroppo solo dalla maggioranza di centrosinistra, un ordine del giorno contro questo decreto sulle fondazioni lirico-sinfoniche: un'iniziativa del gruppo consiliare dell'Italia dei Valori che ha trovato l'appoggio - ripeto - di tutto il centrosinistra. Spero che tale iniziativa possa essere fatta propria anche da altri enti locali, in modo che si levi forte la voce dei territori contro questo provvedimento. Mi spiace che qiestp ordine del giorno non sia stato approvato dagli amici della Lega (ovviamente parlo della Provincia di Torino), perché la Lega, che tanto invoca il federalismo e che quindi tanto dovrebbe avere a cuore,

dei tagli in modo orizzontale, senza avere alcuna attenzione (diversamente da quello che il Ministro oggi ci ha detto e che rimane nelle sue parole, ma non nei fatti e nei contenuti di questo provvedimento) appunto alle realtà territoriali importanti che producono cultura. Potrei citare, per campanilismo, il Teatro Regio, ma è già stato detto molto bene anche da altri colleghi - tutte le nostre realtà delle fondazioni lirico-sinfoniche meritano attenzione.

ma in realtà è un provvedimento che ancora una volta porta l'impronta pesante del ministro Tremonti, come peraltro tutti i provvedimenti che questo Governo e questa maggioranza stanno portando avanti sui temi dell'università e della scuola, dimostrando quindi sostanzialmente una scarsissima attenzione a quello che il mondo della cultura offre, e cioè la formazione ed il senso civico dei cittadini.

significativamente dato un contributo importante di discussione per migliorare questo testo, ed effettivamente alcuni miglioramenti sono stati apportati, ma non ovviamente tutti quelli che ci si sarebbe aspettati.

probabile che attraverso un confronto serratissimo (anche il Gruppo dell'Italia dei Valori ha interesse ad arrivare ad una riforma, ma ad una riforma vera, significativa di questo settore) forse un disegno di legge consentirebbe di apportare quei miglioramenti che fino ad oggi in questo decreto-legge non sono contenuti. Quello che spiace poi di questo provvedimento è che

secondo la quale, così come proposta dal Governo, si sarebbe dovuto prevedere un taglio del 50 per cento delle risorse integrative qualora non si fosse arrivati al rinnovo entro un anno

alla firma del contratto ed in ogni caso al massimo un 5 per cento di riduzione della retribuzione integrativa. Ciò che questo provvedimento a mio parere ha nel suo DNA (e quindi si capisce che è un provvedimento che nelle sue linee guida è stato dettato dal ministro Tremonti e non dal ministro Bondi), è che, anziché che, anziché sostenere una razionalizzazione, una migliore organizzazione e - perché no? - un miglior funzionamento delle fondazioni lirico-sinfoniche, e anche e soprattutto, come spesso il Ministro nei suoi interventi anche pubblici ha ricordato, una incentivazione all'apporto di capitali privati, in realtà ha appuntato la sua attenzione unicamente sui lavoratori, indicando i poveri lavoratori del comparto come colpevoli, o quasi, del dissesto finanziario delle fondazioni lirico-sinfoniche, e peraltro accomunando tutte le fondazioni in un unico, grande pentolone. Investire nella cultura

così altamente specializzato e specialistico, non sono soldi buttati via, perché investiti nella cultura. Un Paese che rinuncia ad investire nella cultura, a a mio modestissimo parere, non ha futuro. Tra l'altro, la nostra Italia è una Nazione che ha una grande tradizione culturale. Sarebbe, dunque, un peccato se uno dei settori che rappresenta una delle grandi eccellenze del nostro Paese venisse penalizzato in questo modo. Per allestire uno spettacolo - lo sappiamo tutti, ma è bene ricordarlo - ci vogliono tecnici, artigiani e professionisti con provata e altissima professionalità ed esperienza in un numero idoneo a sostenere le grandi produzioni che le nostre fondazioni lirico-sinfoniche portano avanti.

in sede emendativa in quest'Aula, di rivedere ancora tutte quelle parti del provvedimento che non pongono

di considerare il problema dei lavoratori di questo comparto, che non meritano di essere penalizzati, perché sono una grande risorsa per il nostro Paese. Signor Presidente, rappresentanti del Governo, colleghi senatori, intervenendo in Commissione sul decreto per le fondazioni lirico-sinfoniche mi sono permesso di ricordare la risoluzione sull'argomento del 18 marzo 2009 della quale sono stato uno dei due relatori. Nell'occasione tutti i membri della Commissione si erano trovati concordi nel sottoscrivere alcuni punti fondamentali. Fra gli impegni del Governo, a parte l'adeguamento del FUS e gli incentivi per una significativa contribuzione da parte degli enti locali, si prevedeva l'adozione di iniziative volte a favorire una maggiore stabilità del settore tramite strumenti di finanziamento a carattere pluriennale per permettere di conoscere con il giusto anticipo le risorse di cui disporre al fine di mettere in atto una corretta gestione delle stesse. Questo è un punto rilevante per assicurare una buona programmazione dei lavori alle fondazioni ed è opportuno quindi avere un preciso riferimento al riguardo nel provvedimento che stiamo esaminando. del finanziamento, sono fondamentali le agevolazioni fiscali e gli incentivi ai contributi da parte dei soggetti privati. Questo aspetto, presente nella risoluzione, mi sembra cruciale per incrementare la produttività delle fondazioni. È evidente che i finanziamenti statali, pur indispensabili, non possono essere l'unica fonte di finanziamento da cui far dipendere la sopravvivenza delle fondazioni. È necessario un investimento da parte degli enti locali e dei privati che possa supportare il buon andamento dell'attività culturale. Il contributo dello Stato è insostituibile, ma la stessa natura giuridica delle fondazioni impone l'approvvigionamento di risorse da parte di *sponsor* e privati. Esistono forme di agevolazione finanziaria utilizzate in altri settori dello spettacolo, come per esempio il cinema. La partecipazione e privati contribuisce inoltre ad avvicinare la cultura lirica al grande pubblico, rafforzando il legame identitario fra cultura e territorio. Un altro punto da sottolineare è quello relativo alla responsabilità della gestione delle fondazioni. Nella risoluzione, fra gli impegni, era contemplata la richiesta alle fondazioni lirico-sinfoniche di inserire con chiarezza negli istituti che è attribuita all'amministratore generale, ovvero sovrintendente, la responsabilità della gestione (che dovrà rispondere alle linee di indirizzo e di bilancio disposte dal consiglio di amministrazione) nonché l'adeguata autonomia decisionale. Devo riconoscere che l'approvazione in Commissione del nostro emendamento 1.100 (testo 2) riafferma in parte tali principi, anche se il fatto che talune disposizioni siano state espunte in quanto presentano difficoltà di ordine finanziario non ci consente di dichiararci del tutto soddisfatti.

A tal proposito, voglio richiamare l'attenzione sul lavoro sviluppato dalla 7a Commissione in materia cinematografica a partire dai disegni di legge presentati dal Popolo della Libertà e dal Partito Democratico, fra loro analoghi, cui si è successivamente aggiunta la proposta innovativa, di ispirazione federalista, della Lega Nord, cioè il disegno di legge n. 1422, a prima firma del senatore Luciano Cagnin. Ci auguriamo che, evitato il rischio di affrontare frettolosamente l'argomento nell'ambito di questo decreto-legge,

*(PdL)*. Signor Presidente, in effetti sono giorni in cui il mondo della cultura e dello spettacolo in Italia è al centro dell'attenzione della nostra attività legislativa, prima con il decreto che stiamo discutendo in quest'Aula e poi con i tagli previsti dalla manovra economica del Governo del ministro Tremonti. Io penso che quello culturale sia il più grande patrimonio di questo Paese:

Nelle arti figurative, nella letteratura, negli studi sulla nostra storia e politica (e penso in questo caso alle celebrazioni per il 150º anno dell'unità del Paese), ma anche nella musica, nello spettacolo e nello sport l'Italia rappresenta per tutti un modello da seguire e da rispettare. Dico, queste parole perché fin troppo spesso, all'orgoglio per la nostra Nazione e per i risultati che noi italiani sappiamo conseguire, subentra una visione negativa di noi e del nostro modo di rapportarci alle altre grandi Nazioni europee, e non solo. Ci sono molti tra di noi che amano ridicolizzare il nostro Paese agli occhi della stampa estera, fornendo un'immagine caricaturale che mi chiedo a chi possa giovare: all'Italia, al nostro Paese, no di certo. Purtroppo, non stiamo vivendo una fase di espansione della nostra economia: è una realtà che, nonostante le parole dei colleghi dell'opposizione che vorrebbero fare credere ai cittadini che siamo solo noi gli sfortunati - accomuna da oltre un anno tutto il mondo occidentale. Illustri economisti la hanno più volte definita la crisi più grave di sempre, dopo quella del 1929. Abbiamo visto cosa è successo in Grecia e cosa potrebbe succedere altrove, dove il rischio del collasso è dietro l'angolo. La Spagna del tanto decantato Zapatero viaggia alla media di un disoccupato ogni cinque persone, mentre anche il neoeletto Governo inglese ha annunciato anni di sacrifici per il popolo britannico. E che dire della Germania, tradizionale locomotiva economica d'Europa, che ha appena varato una manovra economica che prevede un taglio di 80 miliardi di euro fino al 2014? Fortunatamente l'abilità del ministro Tremonti e la coesione del Governo hanno fatto sì che la crisi non abbia toccato il nostro Paese in modo così duro come altri, vittime anche della speculazione finanziaria.

ha come obiettivo la riforma del settore sulla base dei principi di efficienza, economicità e imprenditorialità, per rendere il più funzionale possibile degli enti la cui crisi si è protratta nel corso degli anni. una riforma che è stata richiesta da anni dagli stessi amministratori di queste società e dai loro stessi dipendenti. Certo, fare cultura costa tanto, anche allo Stato che deve predisporre finanziamenti. Si calcola che le 14 fondazioni liriche del nostro Paese assorbano circa il 50 per cento dei finanziamenti pubblici del settore, per le spese di mantenimento e quelle relative alle oltre 5.000 persone che vi lavorano. Una più corretta e razionale ripartizione delle risorse è non solo benvenuta, ma anche necessaria. Vorrei però che non si considerassero i lavoratori di questo settore come di serie B, o minori rispetto a quelli delle aziende o delle fabbriche. Un posto di lavoro perso è e rimane sempre tale, che sia in un teatro o a Termini Imerese. Spesso la riqualificazione del personale che lavora in questi enti è difficile tanto quanto quella degli operai delle fabbriche dismesse; se ci saranno dei tagli, dolorosissimi, sarà importante che lo Stato non faccia sentire solo e abbandonato al suo destino chi ne è stato vittima e non lasci indietro nessuno. Un discorso a parte merita - a mio avviso - una delle grandi istituzioni culturali del nostro Paese, il Teatro alla Scala di Milano. Nel 2009 la Scala ha chiuso il bilancio in maniera nuovamente positiva, con la presentazione di un utile di 40.000 euro, modesto ma corretto in relazione alla natura della Fondazione e alla sua missione, la quale non è orientata al *surplus* economico economico ma a produrre cultura, nel rispetto dell'equilibrio tra costi e ricavi. Il teatro non è riuscito solamente a coprire i costi, ma anche ad aumentare la sua attività produttiva, portando il numero degli spettacoli, dal 2004 ad oggi, da 200 a 319 e le *tournée* fuori sede in Italia e all'estero a 47. Queste rappresentazioni sono state rese possibili dal *budget* di 124,5 milioni e da un patrimonio netto attestatosi intorno ai 35 milioni. Di questo vanno fatti i complimenti al sovrintendente Stéphane Lissner che, con competenza e serietà, ha portato il teatro ad eccellere. Ci vuole un occhio di riguardo nel trattamento della Scala, la quale non può essere messa sullo stesso livello dei tanti, troppi carrozzoni mangia finanziamenti statali, sia per il prestigio internazionale del Teatro, sia per la corretta gestione delle risorse che fino a questo momento ha sempre dimostrato. Vale la pena tenere sotto occhio la situazione della Scala, perché non vorrei che, per l'insipienza di qualche scialacquatore, ci finisse di mezzo anche chi non c'entra nulla. Penso che, per dare al mondo della cultura italiana la possibilità di svilupparsi al di fuori delle sovvenzioni statali e al mito della cultura pubblica, ci voglia un programma di defiscalizzazione defiscalizzazione degli investimenti in questo settore. La procedura attuale è certamente migliorabile, ma non incentiva chi è disponibile a versare delle ingenti somme alle fondazioni e alle associazioni. Il mecenatismo in Italia c'è, c'è stato e dovrebbe essere considerato una risorsa fondamentale, specie in una fase storica dove non è possibile supportare la cultura da parte dello Stato, di tutti gli Stati, come una volta. I dati sull'istruzione nel nostro Paese non sono sempre confortanti, per quanto riguarda sia la scolarizzazione che l'accesso all'istruzione stessa da parte dei cittadini. L'Italia dà l'idea di sottovalutare se stessa, quello che può fare per i suoi cittadini e per mettere a disposizione di tutti un patrimonio che non ha eguali in tutto il mondo. La cultura va coltivata, diffusa, insegnata e cercata, ripeto Teniamo presente tutti - maggioranza e opposizione, operatori del settore e artisti - che tutelarla è, prima che una questione politica, una questione di grande civiltà.

a cui purtroppo non è stato dato alcun ascolto, è incostituzionale e lesivo della dignità e della professionalità dei lavoratori. Già è stato detto dai colleghi che mi hanno preceduto nella presentazione delle pregiudiziali: siamo di fronte - come ormai è tradizione di questo Governo e di questa maggioranza ad un decreto palesemente anticostituzionale, mancando - come previsto invece dall'articolo 77 della nostra Costituzione - dei presupposti di necessità e urgenza. A dimostrazione di questo è il fatto che in molti articoli ci troviamo in presenza di misure con effetto negli anni a venire (come nel caso dei regolamenti previsti dall'articolo 1 per la modifica organica della materia lirico-sinfonica il cui termine è di 12 mesi). Tale carenza dei requisiti costituzionali di necessità e di urgenza si sostanzia altresì nel mancato rispetto delle prescrizioni di cui all'articolo 15, comma 3, della legge n. 400 delle 1988, secondo cui i decreti-legge devono contenere misure di immediata applicazione e il loro contenuto deve essere specifico, omogeneo e corrispondente al titolo. Il decreto-legge, in moltissime delle sue parti e indipendentemente dalle norme ad effetti pluriennali ivi contenute, non contiene affatto norme immediatamente applicabili con chiari e circostanziati effetti normativi. Per quanto concordiamo sulla necessità di una riforma della materia, riteniamo sia arrivato il momento di intraprendere un percorso di investimento su una nuova politica culturale e non possiamo accettare che si scarichi sui lavoratori tutto il peso di questo decreto.

la centralizzazione e ripubblicizzazione della contrattazione collettiva nazionale con il trasferimento della funzione di rappresentanza dall'ANFOLS ad una agenzia di fatto governativa quale è l'ARAN (una norma che snatura il carattere delle fondazioni, di fatto trasformandole in istituzioni pubbliche); l'ingerenza nella contrattazione di secondo livello, con la decadenza dall'entrata in vigore del semplice contratto collettivo nazionale di tutte le clausole e gli istituti inerenti i contratti integrativi aziendali frutto degli accordi del 1993, che dovranno essere rinegoziati tra le parti; la decurtazione del trattamento economico aggiuntivo derivante appunto dalla contrattazione integrativa aziendale che, perlomeno - grazie ad un nostro emendamento - è stata ridotta dal 50 per cento al 5 per cento in caso di mancata stipula del contratto nazionale; il prepensionamento dei ballerini, che peraltro si pone in netta controtendenza rispetto all'elevamento dell'età pensionabile di tutte le altre categorie di lavoratori e che comporta comunque delle conseguenze sull'ammontare finale del trattamento di quiescenza loro spettante. Pur essendo stati approvati alcuni emendamenti migliorativi in Commissione, di cui però non conosciamo l'esito in Aula, risultano purtroppo confermate nel testo norme pericolose e antisindacali. L'unico obiettivo del Governo sembra dunque essere quello di penalizzare una categoria, immagino considerata politicamente lontana, con misure vessatorie ed illegittime. Dobbiamo inoltre opporci alla logica dilagante secondo cui la cultura è un bene superfluo e, come tale, in un periodo di crisi come quello attuale, il primo settore a subire dei tagli. Al contrario, riteniamo che il teatro e la cultura abbiano un ruolo civile e sociale indispensabile, oltre che essere comunque una voce della nostra economia e comunque di un comparto di lavoratori e relative famiglie che il nostro Paese non può ignorare. Purtroppo non possiamo non leggere una coerenza di governo in tutti questi tagli indiscriminati che toccano la crescita culturale del nostro Paese: dai tagli alla scuola, all'università e alla ricerca a quelli ai teatri e agli enti lirici fino al bavaglio ai mezzi di informazione con il decreto-legge sulle intercettazioni: un disegno preciso che sembra mirare a fare dei cittadini italiani dei sudditi. Ancora una volta questo Governo opera tagli indiscriminati e, quel che è peggio, in un settore in cui l'Italia è sempre stata *leader* internazionale. Come ha detto in proposito il grande maestro Barenboim, disinvestire nella cultura significa ignorare il patrimonio culturale italiano e lanciare un messaggio negativo a livello di immagine del nostro Paese. quando all'estero si pensa all'Italia, si pensa a Dante, a Michelangelo, ma anche a Giuseppe Verdi. Voglio esprimere, infine, la convinta solidarietà del mio Gruppo, l'Italia dei Valori, ai lavoratori dello spettacolo colpiti da questo sciagurato provvedimento. *(Applausi

se questo decreto serve davvero a riformare le fondazioni lirico-sinfoniche del nostro Paese. È un decreto il cui testo, un po' modificato in Commissione, con un lavoro veramente serio e approfondito, arriva in Aula senza sapere se ciò che

L'articolo 5 è stato soppresso con un emendamento in Commissione. Credo che lei non farà fatica ad accoglierlo, perché in questa sede stiamo facendo la legge quadro sul cinema.

strutture di contorno, sono le persone, sono gli artisti - sia quelli che appaiono sul palcoscenico sia quelli che vi lavorano dietro - i protagonisti. L'arte, nel teatro e nella lirica, è frutto ed è tributaria anche dei sarti, dei coreografi, dei pittori, e si può quindi definire questo, pensare di mantenere posti di lavoro in un momento di crisi significa pensare a qualcosa che è richiesto. Non viviamo in un Paese diverso ed in un'Europa diversa da quella in cui vive lei, signor Ministro, e vivono i nostri colleghi della maggioranza. Questa crisi la conosciamo. Possiamo solo rimpiangere che voi non abbiate avuto il coraggio di dire da subito che sarebbe stata così grave. Ci si è illusi, avete illuso e adesso arrivano pesanti provvedimenti quello al nostro esame. Vorrei chiedere a lei, Ministro, se si sente di tagliare con un colpo di penna una di queste fondazioni, che non sono legate alla territorialità ma ad una tradizione. Non c'è alcuno al mondo che non conosca, non solo la Scala, ma anche l'Arena di Verona, la Fenice, il San Carlo. Questi teatri hanno una loro specificità, che ha riconosciuto anche lei. Pensi all'Accademia di Santa Cecilia di Roma, la più antica, che non fa solo spettacoli lirico-sinfonici, anzi. A Roma poi, capitale d'Italia, c'è anche il Teatro dell'Opera. Abbiamo a che fare, se mi consente, con una imprenditorialità di un capitalismo, che si chiamerebbe

dell'ente potesse corrispondere una capacità di finanziamento diversa, commisurata, proporzionale, di qualsiasi tipo, del sistema pubblico, che puntasse alla valorizzazione. Invece, non abbiamo potuto discutere. C'era una risoluzione che era davvero una linea guida. Avremmo impiegato lo stesso tempo, signor Ministro, anzi, poiché la risoluzione è di un anno precedente, forse a questo punto avremmo avuto già la riforma degli enti lirici. Ma chi glielo fa fare di portare avanti un ragionamento così affrettato? La Camera dei deputati avrà pochissimo tempo per Qui trova il consenso per fare un'operazione importante anche dal punto di vista dell'unità del Paese, degli investimenti, della tutela del posto di lavoro e - mi consenta - di un grande indotto. Può immaginare cosa significhi una stagione breve dell'Arena di Verona rispetto all'indotto per tutta la zona del lago di Garda, o la circostanza che una di queste fondazioni non vada più all'estero. Chissà quante volte i suoi colleghi, addirittura il Primo ministro, a Tokio o a New York, hanno trovato una di queste fondazioni che stavano da veri ambasciatori, una storia, una cultura e una tradizione. In un momento di grande crisi purtroppo il Governo, ma in realtà il commissario di tutti i Ministri, il ministro Tremonti, in essere un provvedimento così abborracciato che ha messo l'Arena di Verona tra le fondazioni da abrogare. Lei ha dovuto riconoscere l'errore ottenendo

Non salvaguardare la cultura significa aumentare il livello di inciviltà. Sono d'accordo con la mia collega Ombretta Colli, che concludendo il suo intervento ha detto che si tratta di un fatto di civiltà.

e coloro che non lo sono debbano essere tagliati fuori dalla cultura? La cultura in generale, non solo la scuola o l'università, elevano il Paese. Abbiamo bisogno che anche i ceti medio-bassi possano apprezzare questa cultura, perché diventeranno migliori loro e difenderanno il Paese, perché questa è la vera materia prima, non ne abbiamo altre. Questo Governo, per superare questo momento ciclico, avrebbe potuto scegliere indirizzi strategici di investimento esattamente nell'immateriale,

questo decreto del ministro Bondi ha il grande merito di affrontare finalmente la storica crisi strutturale delle fondazioni lirico-sinfoniche la cui situazione finanziaria, drammaticamente deficitaria a causa di una struttura dei costi troppo rigida, pesa enormemente sulle risorse a disposizione del Ministero dei beni culturali condizionandone negativamente l'intera politica culturale. È quindi un intervento legislativo, quello del ministro Bondi che, proprio in virtù dell'amore e del rispetto che si deve ad una tradizione artistica, punta a ristrutturare e riordinare con urgenza e senso di responsabilità il settore lirico-sinfonico, onde evitarne il generale collasso. Un collasso annunciato dai numeri che lo stesso Governo fornisce, quando ricorda che dal 2002 al 2008 le 14 fondazioni liriche hanno accumulato perdite per complessivi 200 milioni e passa di euro, a fronte di una situazione patrimoniale che vede eroso anche il loro patrimonio indisponibile, costituito dal diritto d'uso gratuito degli immobili. Il tutto con elevatissimi interessi passivi generati da un continuo ricorso al credito bancario, nonostante la tempestività dell'erogazione di contributi statali; contributi, peraltro, totalmente assorbiti dalle spese di mantenimento e in particolare dalla spesa per il personale, pari a circa il 70 per cento dell'intero finanziamento pubblico. Eppure, dinanzi a dati così eloquenti e ad una rappresentazione oggettiva della crisi del settore e degli interventi necessari ad affrontarla, non vi è stata lo dico con rammarico - una comune assunzione di responsabilità. In sostanza, l'opposizione di centrosinistra ha scelto di voltare le spalle al problema, distogliendo lo sguardo dalle innovazioni e dalle riforme contenute nel decreto-legge, per guardare solo ai tagli, come se i tagli come se i tagli al FUS non rappresentassero la condizione necessaria per rivedere il meccanismo di erogazione dei contributi su base meritocratica, che per la prima volta si è voluto prevedere in un provvedimento di legge. Ma non c'è nulla da fare: l'opposizione di centrosinistra ha voluto voltare la testa per non vedere le indicazioni normative e le regole gestionali che il decreto-legge Bondi detta ai fini di introdurre criteri di correttezza, efficienza ed economicità nell'amministrazione delle fondazioni lirico-sinfoniche. È stata ed è, quella del centrosinistra, una fuga dalla realtà. Eppure, fuggire dalla realtà per rifugiarsi nella comoda retorica del valore assoluto della cultura può forse servire a guadagnarsi il plauso di qualche orchestrale o direttore d'orchestra (il cui *cachet* in Italia è peraltro pagato più che altrove), ma non serve a salvare le fondazioni lirico-sinfoniche dal disastro. È questo il E che senso ha allora parlare sempre astrattamente di cultura, prescindendo da qualsiasi dato o valutazione di carattere economico? Quasi non esistesse un rapporto fra la struttura economica e quella che un autore ormai abbandonato dalla sinistra, come il povero Marx, chiamava la sovrastruttura culturale. Io credo che oggi fare cultura significa anche fare quadrare i conti delle fondazioni lirico-sinfoniche. Per stare quindi sul concreto, senatrice Garavaglia, prendiamo il caso della Fondazione del Maggio che gestisce il Teatro comunale della mia città, Firenze. I proventi da biglietteria coprono appena l'8 per cento del totale delle entrate. Al resto provvede lo Stato attraverso il FUS, con più di 20 milioni di euro, mentre il Comune, la Provincia e la Regione erogano 6 milioni di euro e i pochi privati (da banche e società assicurative, che hanno peraltro ridotto la loro presenza) si fermano a quota 3 milioni di euro circa. fatto il contributo FUS dello Stato e quello degli enti locali serve solo a pagare gli stipendi, che ammontano a 26 milioni di euro l'anno mentre le produzioni sono finanziate dalla biglietteria, da ricavi vari e dai privati per soli 7 milioni È evidente che ciò crea uno squilibrio economico, in base al quale più si fa più si spende, tant'è che il bilancio della Fondazione del Maggio musicale fiorentino è ed è sempre stato in *deficit* passando dai 12 milioni di euro di buco sotto la gestione quadriennale di Merlini, ai 13 milioni e mezzo di euro nei tre anni di Van Straten. Tanto che per salvare il Teatro, nel 2005, il commissario ministeriale dovette provvedere alla vendita del patrimonio immobiliare costituito da un'ex area industriale ceduta dal Comune alla Fondazione. E così, senza patrimonio, il disavanzo si è attestato attorno a 7 milioni e mezzo di euro nei quattro anni di Giambrone, il quale, da buon sovrintendente, è riuscito comunque a ridurre il rosso, fino ad arrivare nel 2009 ad uno sbilancio di 2 milioni, grazie soprattutto al ricorso al blocco del *turnover* che, guarda caso, è uno strumento indicato dal decreto-legge Bondi per diminuire la spesa storica delle fondazioni. Non solo. Il contratto integrativo stipulato dal Teatro fiorentino, composto da oltre dieci voci diverse, vale 4 milioni e mezzo di euro l'anno. Ora, se fosse stato disdettato per il 50 per cento del suo valore, il bilancio della Fondazione avrebbe potuto chiudersi in pareggio, se non addirittura con un lieve attivo,

non dal centrodestra ma da una profonda crisi economico-finanziaria e, nella fattispecie, da una spesa storica fuori controllo del settore lirico-sinfonico. Certo, l'opera va comunque sovvenzionata. E pubblico e privato devono farsene carico perché la musica è parte integrante della nostra identità nazionale. Pertanto, il problema non è perciò se lo Stato deve o no investire, ma come e quanto. Non si può continuare a dare soldi a fondo perduto, sapendo già che i bilanci saranno in rosso. Bisogna cambiare, riequilibrando gli interventi tra pubblico e privato. Il decreto Bondi ha centrato il problema, indicando misure e strumenti concreti: modificare la struttura troppo rigida dei costi di gestione delle fondazioni lirico-sinfoniche e aumentare le risorse esterne dei privati. Questo è e deve essere l'indirizzo generale. Resta pertanto sullo sfondo, proprio per favorire l'ingresso e l'apporto di soci privati, l'esigenza, signor Ministro, di rivedere la sciagurata legge Veltroni, che istituì le fondazioni lirico-sinfoniche senza dotarle di patrimonio e, soprattutto, senza definirne con chiarezza la natura. infatti, possono essere sì considerate persone giuridiche di diritto privato, ma solo fino a un certo punto, tant'è che nei fatti (ripeto, nei fatti) si presentano come organismi di diritto pubblico in quanto, tra l'altro, beneficiarie di finanziamenti pubblici. È una mostruosità giuridica, le cui ambiguità e contraddizioni ostacolano gestioni improntate a criteri di efficienza e imprenditorialità. Senza considerare che tale loro indefinita natura risulta ulteriormente accentuata dal fatto che tutte le fondazioni sono, per statuto, presiedute dai sindaci delle città in cui sorgono, i quali troppo spesso tendono a servirsene come di un podio o a considerarle alla stregua di una semplice società partecipata del loro comune, aumentando così la confusione che regna attualmente sotto il cielo dell'opera italiana.

1a Commissione permanente, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, osservando che, agli articoli 2 e 3, la disciplina ivi prevista, intervenendo in modo eccessivamente dettagliato sull'autonomia negoziale degli enti lirico-sinfonici, in particolare per quanto attiene alla contrattazione collettiva e alla disciplina dei contratti integrativi aziendali, presenta alcuni profili di contrasto con le competenze delle Regioni e degli enti locali in materia». 1a Commissione permanente, esaminati gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo». «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti trasmessi dall'Assemblea e relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza,

le seguenti parole: "con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato". alla proposta 7.0.70, al comma 2, siano soppresse le parole: "e adotta le azioni opportune per restaurare e valorizzare i Luoghi della Memoria nazionale presenti sul territorio italiano". è altresì reso nel presupposto che si proceda nell'ambito delle risorse già previste a legislazione vigente. Esprime, infine, parere non ostativo sulle restanti proposte. Resta sospeso il parere sugli emendamenti 3.65 (testo 2) e 3.154 (testo 2)».

il punto non è quello di accusare il Governo di avercela in particolare con il mondo della lirica e dell'opera: dell'opera: piuttosto, quello di non intervenire con qualche innovazione vera, di sistema, in una difficoltà strutturale che certamente il decreto non affronta se non su alcuni aspetti, peraltro in modo assai discutibile. Anche in questa

Non abbiamo problemi nel portare avanti questo decreto-legge, perché abbiamo i numeri e siamo convinti che

al costo di un magistrato. Nemmeno quello si vuol fare. Ma c'è di più: è ora di rivedere le tante indennità assurde dei contratti integrativi:

Secondo voi, è positivo il fatto che 14 enti lirici abbiano 14 contratti diversi?

garantire un adeguamento delle risorse da destinarsi al FUS tale da permettere il mantenimento in vita del settore; prevedere specifici strumenti di raccordo dell'operato delle fondazioni al fine di realizzare la più ampia sinergia operativa possibile; destinare una quota crescente del finanziamento statale in base alla qualità della produzione; incentivare un'adeguata contribuzione da parte degli enti locali; introdurre adeguate misure per accrescere la produttività del settore; adottare ogni opportuna iniziativa, ove necessario anche a carattere normativo, volta a favorire una maggiore stabilità del settore, tramite strumenti di finanziamento a carattere pluriennale che permettano di conoscere con il giusto anticipo le risorse di cui disporre al fine di mettere in un atto una corretta gestione delle stesse; prendere in considerazione l'opportunità di costituire un tavolo di confronto con le diverse fondazioni ed i rappresentanti sindacali dei lavoratori, al fine di revisionare gli aspetti carenti della riforma attuata con il decreto legislativo n. 367 del 29 giugno 1996; prevedere che il finanziamento dello Stato garantisca almeno il costo del contratto collettivo nazionale di lavoro; richiedere alle fondazioni lirico-sinfoniche che gli statuti attribuiscano con chiarezza all'amministratore generale, ovvero al sovrintendente, la responsabilità della gestione che dovrà rispondere alle linee di indirizzo e di bilancio disposte dal consiglio di amministrazione, nonché l'adeguata autonomia decisionale; prevedere la valorizzazione del sistema dei grandi teatri d'opera italiani, così come definiti dalla legge 14 agosto 1967, n. 800, all'interno di un progetto di riforma che valorizzi le eccellenze specifiche, ripartendo dal principio dell'intervento culturale, inteso come investimento e non come spesa; mantenuta la capacità di produzione culturale sul territorio e il genere di spettacolo (lirica, balletto, musica sinfonica) come tipicità caratterizzanti l'identità ed i fini istituzionali delle fondazioni, assicurando anche, a garanzia della qualità produttiva, la consistenza organica dei complessi stabili, con particolare riguardo a quelli indispensabili alla produzione (professori d'orchestra, artisti del ballo e del coro, maestranze, tecnici di laboratorio e palcoscenico); prevedere la possibilità di specifici finanziamenti statali per le fondazioni con funzione perequativa e premiante, in ragione dei risultati culturali più interessanti sul piano delle proposte, della qualità e dei progetti culturali; mettere in campo ogni azione volta a incentivare l'intervento nel settore dei soggetti privati, garantendo agevolazioni fiscali alla contribuzione privata; valorizzare le finalità e il carattere sociale delle fondazioni lirico-sinfoniche, il loro ruolo educativo verso i giovani, la loro *mission* di trasmissione dei valori civili fondamentali (verso cui del resto sono sempre state orientate le grandi istituzioni teatrali e culturali italiane); prevedere l'attivazione di un percorso che coinvolga tutti i soggetti interessati, quali le Regioni, i Comuni, i sovrintendenti delle fondazioni, le organizzazioni sindacali rappresentative. Queste, in sostanza, sono le cose che avevamo chiesto esattamente un anno fa, quando si è cominciato a mettere mano al provvedimento che abbiamo oggi in discussione. Purtroppo, non tutti questi punti sono stati presi nella dovuta considerazione. Il motivo voi lo sapete: c'è una situazione economica particolare e difficile; bisogna intervenire per rimettere in conti sotto controllo, e le risorse che ci sono, come sapete benissimo, sono limitate. Per cui, se con l'emendamento 1.100 siamo riusciti a riproporre buona parte delle linee guida che ho appena elencato, quattro di questi punti sono stati cassati per intervento della Commissione bilancio, che ha fatto i suoi conti. Un punto di soddisfazione per noi è che si proponga la soppressione

una proposta del Gruppo Lega Nord, di ispirazione federalista, che vorrebbe per la prima volta dare spazio anche alle Regioni in merito al modo di utilizzare i finanziamenti messi a disposizione per il cinema. È una novità della quale bisognerà assolutamente tenere conto, perché

per sé, invito i senatori Segretari a verificare.

**Il Senato non approva**. Sono altresì improponibili tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 9, in quanto tale disposizione disciplina unicamente il momento dell'entrata in vigore del decreto-legge. Passiamo all'esame dell'articolo 1 del Signora Presidente, illustrerò brevemente i numerosi emendamenti all'articolo 1. Signor Ministro, lei ha parlato di una riforma che in questo provvedimento non c'è. L'articolo 1 è l'articolo determinante sulla riforma degli enti lirico-sinfonici, e rinvia, in realtà, a dei regolamenti che il Ministero nei prossimi 12 mesi dovrebbe emanare. La riforma della quale il ministro Bondi ci ha parlato non esiste assolutamente in questo decreto-legge. Noi abbiamo fatto uno sforzo emendativo molto forte anche sull'articolo 1, proprio per dare una serie di contenuti a questo provvedimento che non ha nessun contenuto se non quello del taglio

dei finanziamenti, degli sgravi fiscali, di tutto ciò che servirebbe alle fondazioni lirico-sinfoniche e che voi con pervicacia ci avete impedito di affrontare durante la discussione in Commissione e temo, ahimè, ci impedirete di inserire anche durante questo dibattito in Aula. Proponiamo innanzitutto emendamenti soppressivi perché questo articolo, così com'è, è pessimo e dannoso, ma procediamo anche con emendamenti che offrono un contenuto serio e concreto a questa riforma. Mi auguro che il Governo, il relatore e la maggioranza comprendano quello che stanno facendo, la drammaticità della situazione in cui stanno mettendo le fondazioni lirico-sinfoniche e aderiscano ai nostri emendamenti per dare un serio contributo e un serio contenuto a questo provvedimento.

anche modificando le disposizioni legislative vigenti, attendendosi ai seguenti criteri»; seguono criteri generali. Se approveremo questo articolo, daremo mandato al Governo tramite regolamenti al riassetto complessivo delle norme sulle fondazioni lirico-sinfoniche. Né le Commissioni parlamentari, né quest'Assemblea, né le Regioni avranno modo d'intervenire sul provvedimento entro i prossimi 12 mesi l'emergenza sono testimoniate anche dal fatto che il Governo si prende comodamente i prossimi 12 mesi per provvedere a tali regolamenti!).

è stato approvato il nostro emendamento che proponeva di sopprimere l'intero articolo, proviamo a sopprimere almeno il comma 1, che è quello che dà un'impronta a tutto il provvedimento.

1 lede profondamente l'autonomia delle fondazioni, che per noi è il punto di forza della legge istitutiva delle fondazioni lirico-sinfoniche, e, invece di basarsi sulla premialità, come abbiamo proposto in molti emendamenti,

che propone la soppressione del comma 1 in cui si legge: «Con uno o più regolamenti da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, su proposta del Ministero per i beni e le attività culturali, il Governo provvede alla revisione dell'attuale assetto ordinamentale ed organizzativo delle fondazioni lirico-sinfoniche...» l'emendamento vuole sopprimere questo primo comma perché in esso è disciplinata una marcata opera di

il Governo, cari colleghi, dovrà disciplinare l'intera materia derogando, modificando o abrogando norme di rango primario - questo, cari colleghi, è motivo ulteriore per stigmatizzare l'utilizzo dello strumento del decreto-legge:

Credo che i colleghi dovrebbero essere attenti a valutare ciò, per la stessa tenuta di un meccanismo decisionale che il Governo vuole mettere in campo.

dell'organizzazione e del funzionamento sulla base dei principi di efficienza, corretta gestione, economicità ed imprenditorialità, anche al fine di favorire l'intervento di soggetti pubblici e privati nelle fondazioni". Il presente emendamento è volto a sopprimere questo punto, il primo dei criteri direttivi al quale dovrà ispirarsi il Governo nell'adottare Non è infatti possibile immaginare di razionalizzare l'organizzazione, il funzionamento, la corretta gestione e, addirittura, favorire l'intervento dei privati per il tramite di un regolamento delegato in forza

Questo emendamento, però, come ricordato anche in Commissione, è di assoluto buonsenso, perché introduce il concetto, assai più credibile e equo, di valorizzazione delle professionalità,

Stiamo insistendo sulla lettera *a)* perché è paradossale che, in un provvedimento che riguarda le fondazioni lirico-musicali, quando si stabiliscono i criteri ai quali il Ministro deve ispirarsi per emanare i regolamenti il criterio più importante sia quello ed esclusivamente quello della razionalizzazione dell'organizzazione in base a efficienza, corretta gestione, economicità ed imprenditorialità. Non c'è nessun riferimento a quella che dovrebbe essere la missione naturale di una fondazione lirico musicale, cioè la produzione culturale. È stato tra l'altro bocciato appena ora l'emendamento a prima firma del senatore Vita, che faceva riferimento proprio alla valorizzazione delle professionalità. Noi Noi proponiamo di inserire come comma aggiuntivo almeno un riferimento alla valorizzazione del sistema dei grandi teatri d'opera italiani che caratterizzano, come abbiamo detto molte volte, la nostra storia e la nostra

Peccato che in questo provvedimento non si preveda un articolo sulle agevolazioni fiscali. Quindi, diventa difficile commentare un provvedimento. Mi rivolgo ancora al Ministro,

in cui l'articolo 1 è stato formulato. Uno dei criteri previsti per i regolamenti che il Ministero dovrà emanare per cambiare la normativa sugli enti lirico-sinfonici è il criterio eventuale previsione di forme organizzative speciali per le fondazioni lirico-sinfoniche in relazione alla loro peculiarità, alla loro assoluta rilevanza internazionale, alle loro eccezionali capacità produttive,

una gerarchizzazione dei teatri, ovvero l'indicazione di teatri di serie A e di serie B. Siccome non sono proprio sicura che tale ipotesi sia totalmente tramontata, vorrei sottolineare con altrettanta chiarezza che sarebbero inaccettabili decisioni centralistiche, burocratiche e lesive della pari dignità dei teatri italiani. Non esistono teatri di serie A e di serie B, né esistono pubblici di serie A e di serie B ai quali, se mai, offrire spettacoli di ripiego. Voglio dire che il teatro San Carlo non è certo da meno dell'Accademia di Santa Cecilia, né il pubblico del Teatro alla Scala meriterebbe di più del pubblico del San Carlo di Napoli. La qualità deve e dovrà essere garantita a tutti. È per questo che ho presentato questo emendamento, che tende appunto a definire dei criteri, al di là di quello del reddito del botteghino, che facciano la qualità e che vengano veramente messi al centro dei decreti legislativi cui rinvia tale decreto, che probabilmente il Parlamento non potrà mai discutere. Per questi motivi invito a sostenere e a votare l'emendamento

Grazie, signor Presidente. volevo richiamare la sua attenzione su una comunicazione, molto burocratica, che abbiamo trovato stamattina sulle nostre scrivanie, con la quale ci viene comunicato dal Servizio di questura e del cerimoniale che, d'ora in poi, i nostri uffici ci saranno interdetti a partire delle ore 21.

possiamo cavarcela da soli; ci date le chiavi e rimaniamo in ufficio, ma dateci la possibilità di lavorare.

purtroppo ne parliamo del passato - un grande sindaco, che ha ben operato nella nostra Provincia. È sempre stata vicina alle esigenze dei propri cittadini, con fermezza e schiettezza, il che l'ha fatta apprezzare in tutti gli anni del suo mandato. Noi la ricordiamo con stima, e sinceramente credo che tutti i cittadini della Provincia di Treviso, e non solo quelli del suo Comune, Villorba, la ricorderanno per sempre per i suoi grandi meriti. *(Applausi *(PD)*. Signor Presidente, volevo intervenire sullo stesso problema della chiusura degli uffici. Addirittura, per quanto riguarda la Commissione d'inchiesta sul Servizio sanitario nazionale,

Presidente, mi dispiace, ma vorrei intervenire anch'io sullo stesso argomento. Ci troviamo in condizioni veramente difficili di lavoro, spesso con la necessità di predisporre degli emendamenti che devono essere presentati per la mattina successiva, con la necessità di studiare per più Commissioni. Probabilmente questi provvedimenti sarebbero adeguati per il Senato del passato, non per un Senato moderno in cui i senatori sono i primi ad applicarsi sui provvedimenti legislativi in relazione alle loro specifiche competenze. È quindi veramente inammissibile. Ho avuto più volte questioni

e di non dare seguito a questioni di questo tipo. Questo limita la nostra attività, perché siamo impegnati dalle Commissioni per tutta la settimana, poi ritorniamo nei nostri collegi, quindi abbiamo diritto di lavorare e vogliamo lavorare bene. Credo che lei su questo punto debba intervenire. Personalmente sono d'accordo con il senatore del consegnateci le chiavi; noi a questo punto siamo in grado di gestirci da soli, abbiamo risolto la situazione, ma non impediteci di lavorare, perché questo non è possibile.